Oggi con emozione e orgoglio sono al vostro cospetto per illustrarvi i contenuti della relazione annuale sull'amministrazione della giustizia. Emozione, in quanto per, la prima volta, ho l'onore di presentare in quest'Aula la relazione annuale; orgoglio, perché confido di dar conto dei primi importanti risultati ottenuti dal Ministero della giustizia, che rappresentano le fondamenta per una complessiva revisione del sistema giustizia da sviluppare e portare a compimento nel corso della legislatura. Vorrei evidenziare che nel contratto di Governo del cambiamento è stata indicata - quale stella polare del settore giustizia - la necessità di riportare il cittadino al centro del sistema giudiziario. Tale innovativa prospettiva è stata accompagnata da una differente impostazione metodologica, incentrata sull'ascolto, sul dialogo e sulla collaborazione. La costruzione effettiva di una giustizia a misura di cittadino richiede la costante partecipazione al processo di rinnovamento da parte di tutti i soggetti che, a vario titolo, gravitano intorno all'universo giudiziario. Adottando un criterio dialogico e dialettico, si è deciso di intraprendere un'interlocuzione trasversale che coinvolga non soltanto le diverse forze parlamentari, ma anche gli operatori del diritto: magistrati, personale amministrativo, avvocati, gli organismi forensi nonché i fruitori ultimi del servizio, i cittadini, al fine di dar vita a percorsi di riforma condivisi nell'ottica del perseguimento di un miglioramento complessivo dei sistemi di giustizia. Il settore della giustizia rappresenta uno dei pilastri più importanti per un ordinamento giuridico che ambisca a definirsi realmente democratico, e influenza in maniera decisa altri settori strategici, quale quello sociale ed economico. È per queste essenziali ragioni che l'azione ministeriale

che ben si dovesse coniugare con le linee guida contenute nel contratto di Governo del cambiamento. Ritengo, in questo primo inizio di legislatura, di aver fornito dimostrazione di tale apertura, avendo, da un lato, garantito l'indispensabile continuità burocratica propria della pubblica amministrazione, e, dall'altro lato, avendo dato corso - nei limiti della compatibilità politica - a procedimenti legislativi che erano già stati avviati nel corso della precedente legislatura. Il mio auspicio è che in tal modo possa inaugurarsi una stagione di riforme condivise che, pur nel rispetto delle differenze politiche e degli assetti parlamentari, siano condotte nell'esclusivo interesse del Paese, frutto di un sano confronto dialettico e non di uno scontro politico sterile e dannoso, nella responsabile consapevolezza che la giustizia sia un valore e che rappresenti la principale forma di tutela per ogni cittadino che aspiri legittimamente a vedere tutelati i propri diritti. Tanto più è necessario un intervento complessivo se consideriamo come le aspirazioni legittime dei cittadini progressivamente stiano denotando un netto arretramento. Costosa, lenta, incapace di garantire la tutela dei diritti: è questo il giudizio pesantissimo che gli italiani danno alla giustizia nel rapporto Censis 2018. Un terzo della popolazione adulta, il 30,7 cento, vale a dire 15,6 milioni di persone, negli ultimi due anni ha infatti rinunciato a intraprendere un'azione giudiziaria volta a far valere un proprio diritto: un comportamento diffuso trasversalmente in tutta la popolazione ma più forte al Sud, dove raggiunge il 37,5 per cento. Le ragioni possono essere diverse:

denominatore è la costante crescita della sfiducia: sette italiani su dieci pensano che il sistema giudiziario non sia idoneo a garantire pienamente la tutela dei diritti fondamentali dell'individuo. Voglio chiarire che questa sfiducia rappresenta un vero e proprio paradosso se consideriamo che la magistratura e l'avvocatura italiana sono eccellenze a livello internazionale. pertanto, che adesso sia la politica a dover dare nelle sedi istituzionali una risposta ai cittadini sulla loro domanda di giustizia. Mi accingo allora a illustrarvi gli aspetti principali delle innovazioni introdotte nell'anno 2018 e i profili di maggiore interesse del complessivo intervento sulla macchina amministrativa relativa al comparto giustizia, rinviandovi all'integrale lettura della esaustiva documentazione sullo stato della giustizia che ho depositato oggi, per quanto non espressamente riportato in questa sede. Il presupposto fondamentale sul quale è stata improntata l'azione amministrativa è rappresentato dalla convinzione che qualsiasi tentativo di innovazione legislativa risulterebbe inefficace in concreto se non accompagnato e sostenuto da adeguati strumenti organizzativi e dalle necessarie risorse umane e materiali. Le somme destinate alle spese di giustizia sono state fortemente incrementate rispetto al passato considerando che il bilancio di previsione per il 2019 nell'area giustizia prevede un importo di 8.582.653.608 euro, con un aumento rispetto al bilancio di previsione del precedente Governo per il 2018 di oltre 324 milioni. Oggi possiamo dire che la giustizia, alla luce della legge di bilancio appena approvata, rappresenta una vera e propria priorità per questo Paese. è stata rivolta alla problematica della carenza di personale di magistratura e amministrativo attraverso investimenti strutturali e adeguati stanziamenti in bilancio. Si è dovuta fronteggiare, operando una vera e propria inversione di marcia, una condizione di grave scopertura degli organici, frutto di anni di *spending review*. Trattasi di investimenti non episodici, ma sistematici, che sono stati e saranno accompagnati nel prossimo triennio dalla programmazione delle future assunzioni e dalla revisione delle piante organiche in ampliamento, ormai in larga parte inadeguate a causa delle politiche inerziali dell'ultimo ventennio. Un significativo impegno è stato profuso dal Ministero della giustizia nella gestione degli organici della magistratura e del funzionamento degli uffici giudiziari tradottosi nello studio e nell'adozione di misure finalizzate a realizzare una più efficiente distribuzione e allocazione nelle sedi giudiziarie delle risorse di organico disponibili. L'intervento inciderà sugli organici della magistratura attraverso la variazione in aumento delle piante organiche degli uffici garantendo, al contempo, il mantenimento dell'attuale percentuale di copertura degli organici effettivi. Sotto il primo profilo, in attuazione delle linee programmatiche dell'amministrazione della giustizia, all'interno della legge di bilancio è stato previsto l'aumento del ruolo organico della magistratura ordinaria di complessivi 600 magistrati, 530 dei quali con funzioni giudicanti e requirenti di merito, 65 con funzioni giudicanti

limiti delle autorizzazioni di spesa previste nel bilancio di previsione per l'anno 2019 e per il triennio 2019-2021 pari a 90,70 milioni di euro nel triennio. Per quanto concerne la copertura degli organici è stata condotta un'intensa attività di reclutamento attraverso l'indizione, con il decreto ministeriale del 10 ottobre 2018, di un nuovo concorso a 330 posti di magistrato ordinario che, unitamente alla prossima conclusione dei precedenti concorsi indetti rispettivamente con il decreto ministeriale del 19 ottobre 2016 e del 31 maggio 2017, 2017, garantisce la necessaria continuità nell'assunzione del personale attraverso la cadenzata e costante previsione di almeno un concorso all'anno. Al fine di consentire l'assunzione dei magistrati ordinari vincitori di concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della legge di bilancio pari a 360 unità sono state previste maggiori risorse per 84,4 milioni di euro nel triennio 2019-2021. Nel dar conto di quanto il Ministero della giustizia nel corso della precedente legislatura ha disposto in tema di magistratura onoraria, ovvero una procedura culminata con la nota del 27 aprile 2018 contenente la proposta di determinazione delle nuove piante organiche degli uffici del giudice di pace e degli uffici di collaborazione del procuratore della Repubblica, si sottolinea l'intenzione di questo Dicastero di riconoscere che la stessa magistratura onoraria costituisce una imprescindibile componente nel sistema giustizia. Si precisa che, allo stato, sono allo studio possibili iniziative volte a rendere più efficienti ed equi gli interventi in tema anche e soprattutto attraverso

ha coinvolto sia l'aspetto quantitativo che quello qualitativo, dovendosi al contempo far fronte alla carenza di personale e alla necessità di fornire l'adeguato aggiornamento professionale agli operatori. Per corrispondere all'indifferibile e prioritaria necessità di copertura delle carenze di organico del personale amministrativo, non solo sono stati assunti i vincitori del concorso per assistenti giudiziari in numero di 800, ma si è provveduto allo scorrimento della graduatoria dei candidati idonei che ha portato all'assunzione di ulteriori 2.044 unità le quali hanno preso servizio tra il 9 febbraio e il 19 settembre 2018, ripartite tra gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione giudiziaria. Sono stati inoltre reclutati 131 funzionari giudiziari e 13 dirigenti di seconda fascia che hanno sottoscritto il contratto individuale di lavoro il 2 ottobre scorso, oltre alle ultime assunzioni nell'ambito delle categorie protette. Con la legge di bilancio sono state inoltre previste maggiori risorse per 224,77 milioni di euro nel triennio 2019-2021 in vista dell'assunzione a tempo indeterminato di 3.000 unità di personale amministrativo giudiziario della terza e della seconda area funzionale, di cui 97 unità di personale per giustizia minorile e di comunità di cui viene incrementata la dotazione organica della carriera dirigenziale di sette unità. Parimenti, per il personale tecnico-amministrativo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, si è prevista l'assunzione a tempo indeterminato di 260 unità della terza e seconda area, nonché di 35 dirigenti di istituto penitenziario. Si tratta di un primo grande passo per permettere agli uffici giudiziari di recuperare efficienza, messa in crisi dalle cessazioni dal servizio non compensate da un adeguato *turnover*, primo passo che ha consentito di passare da una scopertura di organico nazionale al 31 dicembre 2017

concorsi pubblici per allievo agente per complessivi 1.438 posti con assunzione dei vincitori nei mesi di novembre e dicembre 2018. Inoltre, nel corso del 2018, 1.331 allievi agenti hanno frequentato e terminato il corso di formazione con l'immissione in servizio e 977 unità di personale, selezionate con concorso interno, sono state avviate al corso di formazione per la nomina della qualifica di vice ispettore del Corpo la cui conclusione è prevista nel mese di marzo 2019. Quanto al personale amministrativo, sono perfettamente consapevole delle aspettative che ci sono per quanto riguarda lo scorrimento della graduatoria a tutt'oggi esistente. In tal senso, mi preme dire che, dopo aver effettuato con la legge di bilancio un'iniezione quantitativa di risorse,

sulle velocizzazioni delle procedure, consentissero concretamente di perseguire l'obiettivo primario di collocare il cittadino, fruitore del servizio giustizia, al centro del sistema. Per tali ragioni, l'azione del mio Dicastero nel 2018 è stata focalizzata sulle procedure di valutazione dei risultati e su quelle di trasparenza. Come ho anticipato, la fissazione di obiettivi chiari, specifici e misurabili risponde a un duplice scopo, in quanto è indispensabile, da un lato, per una corretta comparazione della rispondenza tra risultati

tutte le articolazioni ministeriali e l'organismo indipendente di valutazione. Anche l'attività svolta dall'ispettorato generale, coerentemente con gli obiettivi e le linee guida dell'azione ministeriale, si è caratterizzata non solo quale attività di mero controllo della regolarità degli uffici giudiziari, ma soprattutto quale verifica trasparente delle relative *performance,* al fine di offrire un supporto in termini di efficienza e regolarità degli uffici. In siffatta prospettiva, nel corso dell'attività ispettiva espletata nel 2018 si è prestata particolare attenzione al profilo dell'effettività dell'azione giudiziaria connessa alla definitività della decisione e alla sua concreta esecuzione. Tramite ricorso a a prescrizioni, raccomandazioni e rilievi si è data particolare considerazione alle irregolarità o alle lacune che più direttamente incidono sulla qualità del servizio. Le verifiche effettuate si sono concretate quindi nel settore civile sul rispetto della ragionevole durata dei procedimenti, attraverso la gestione dei ruoli e la tempistica dei depositi e sul numero delle impugnazioni, laddove invece nel settore penale l'attenzione è stata diretta soprattutto alla verifica dell'incidenza della prescrizione, delle modalità

di giustizia. Su questo punto tengo a dire che, consapevole del livello altissimo di professionalità della nostra magistratura, che è la migliore in Europa e sicuramente una delle migliori a livello internazionale, proprio nel rispetto di quell'altissimo livello di professionalità, ho ritenuto di dare sempre maggiore impulso all'ispettorato affinché individuasse chi, all'interno di una categoria di livello altissimo - lo ribadisco -, non lavora come dovrebbe, non rispettando prima di tutto i propri colleghi, arrecando un danno al servizio giustizia e, quindi, ai cittadini. La riforma della geografia giudiziaria del 2014, se da un lato ha consentito una

e ha segnato una vera ferita per molte realtà locali, essendo venuto meno un presidio di legalità e sicurezza rappresentato dall'ufficio giudiziario. L'idea di giustizia che si vuole restituire ai cittadini è quella di un bene presente sul territorio, in modo da venire incontro all'esigenza, avvertita specialmente dalle fasce deboli e soprattutto nelle zone fortemente delocalizzate rispetto a quelle dove hanno sede gli uffici, di poter ottenere tutela dei diritti accedendo ad un unico luogo ove convergono gli che, a diverso titolo, partecipano alla costruzione del sistema delle tutele. Questa è la visione che ha ispirato il progetto degli uffici di prossimità,

necessariamente recare presso gli uffici giudiziari. Si tratta di un progetto strutturale su larga scala, che prevede la possibile apertura, grazie alla sinergia tra istituzioni a livello nazionale, regionale e locale, di 1.000 uffici di prossimità, con una dotazione finanziaria di 36.764.941 euro. Gli uffici di prossimità potranno garantire un servizio completo e integrato di orientamento e consulenza, specialmente alle fasce più deboli, per la trasmissione degli atti che non richiedono l'ausilio di un legale, quali ricorsi, istanze, allegati e c'è troppo brusio in Aula. su questioni che riguardano la loro sfera familiare e personale. Mi preme dire che, in passato e chiaramente nella scorsa legislatura, ero stato molto

territorialmente più periferici o comunque in zone in cui il presidio di legalità rimane fondamentale. Ci tengo a dire che, in questo senso, stiamo facendo un monitoraggio attento e sappiamo che la ferita è ancora molto aperta tra i cittadini: questo dà il senso dell'importanza che la la giustizia ha per i cittadini stessi. Sappiamo che gli uffici di prossimità non hanno un collegamento diretto con la geografia giudiziaria, perché sono ben altra cosa, ma sappiamo anche che essi rappresentano un segnale di vicinanza che, esplicandosi nell'ambito della volontaria giurisdizione, in qualche modo avvicina avvicina la giustizia alle fasce deboli della popolazione. L'edilizia giudiziaria è un tema nevralgico, rivestendo un duplice significato: sostanziale e simbolico. È paradossale pensare che i luoghi in cui si amministra la giustizia siano essi stessi fonte di violazione dei diritti dei cittadini, nella loro veste di lavoratori. Uno Stato di diritto non può e non deve consentire simili abusi. L'ossequio agli articoli 3 e 35 della Costituzione impone di creare le condizioni affinché i luoghi in cui si

Al fine di strutturare un programma di interventi organico e da svilupparsi lungo differenti direttrici, è inoltre apparso necessario - e i tragici eventi di questi ultimi giorni lo confermano drammaticamente - avviare una mappatura dell'attuale edilizia giudiziaria, per comprendere la composizione, le criticità e il livello di urgenza degli interventi, sia strutturali, sia di mero adeguamento. Le principali direttrici lungo le quali si è mossa l'attività del Ministero innanzitutto, il recupero dell'immediatezza degli interventi programmati e la tempestività degli interventi di manutenzione degli uffici richiedenti, per i quali le risorse impiegate sono state imponenti e rendono atto dell'attenzione posta dal Ministero alla delicatezza del tema. L'importo per le opere di adeguamento al testo unico (decreto legislativo

il cui dato è particolarmente elevato, essendo pari a 380 contratti per oltre 300 immobili, che costituiscono un capitolo di spesa costante e antieconomico. Il censimento di tali immobili è stato propedeutico alla ricerca di soluzioni alternative, attraverso l'implementazione di indagini di mercato finalizzate alla ricerca di nuovi immobili adeguati rispetto alle esigenze delle strutture territoriali e idonei a interrompere una spesa superflua in capo al Ministero. Risultano allo stato in corso undici indagini di mercato, che riguardano le sedi di Foggia, Catania (dove ci sono due indagini in corso), Modena, Udine, Latina, Benevento, Pistoia, Venezia, Messina, Civitavecchia e Tivoli. il riutilizzo di immobili demaniali aventi una differente destinazione originaria, supportato anche tramite la predisposizione di modelli innovativi di gestione. Attraverso la stipula di protocolli d'intesa (ben nove nel corso dell'anno 2018) con la Cassa depositi e prestiti e l'Agenzia nazionale del demanio, è stato possibile

procedendo alla consequenziale dismissione delle locazioni passive in atto dei rispettivi uffici giudiziari. Parimenti, sono stati individuati immobili di proprietà pubblica in disuso da molti anni, da riqualificare e destinare a usi giudiziari. Menzione a parte merita la risoluzione della nota vicenda riguardante il polo penale del tribunale di Bari, segno tangibile del grado di emergenza e di urgenza cui è giunta la problematica dell'edilizia giudiziaria. La procedura è stata definita in tempi estremamente e oggettivamente brevissimi *(Applausi in locazione dell'immobile sito in Bari, via Dioguardi n. 1, per le necessità degli uffici giudiziari baresi precedentemente allocati nel palazzo di giustizia di via Nazariantz: il tutto senza ricorrere ad alcuna opera di commissariamento. L'Amministrazione ha profuso un impegno incessante nell'attività di ricerca della nuova sede in tempi contingentati, resi ancor più ridotti dalla complessità dell'indagine da svolgere, considerata la quantità degli uffici, di risorse e di personale da allocare. Chiaramente stiamo parlando di una soluzione non definitiva, ma a tutt'oggi stabile.

personalmente sul posto e, con gli uffici giudiziari, abbiamo proseguito (non avviato) un'interlocuzione per gestire al meglio le richieste di sicurezza dei tribunali. L'aumento della funzionalità dei servizi ha connotato anche l'attività di gestione e adeguamento del patrimonio immobiliare destinato al settore della giustizia minorile e di comunità. Gli interventi si sono pertanto incentrati sulla razionalizzazione degli spazi, sull'elevazione degli *standard* di igiene e sicurezza, sull'introduzione di sistemi tecnologici avanzati avanzati per l'ottimizzazione delle attività di controllo e gestione degli istituti penali, nella consapevolezza che l'esecuzione penale nei confronti dei minori manifesta una peculiare necessità di territorializzazione della pena, giacché la rieducazione dei minori deve avvenire integrando il supporto statuale con quello familiare.

ineludibilmente attraverso un'adeguata allocazione di nuove risorse e un'ottimizzazione di quelle esistenti. La vera sfida è rappresentata dalla capacità di contenere la spesa e, al contempo, elevare gli *standard* qualitativi dei servizi offerti all'utenza. Un ulteriore positivo intervento effettuato nell'anno 2018 dal Ministero, per il contenimento e la razionalizzazione

e telematizzazione dei procedimenti giudiziari, con l'avvio del Portale dei servizi telematici, delle notifiche telematiche del giudice di pace entro giugno 2019 e della digitalizzazione in Cassazione. Entro il 2019 si raggiungerà la prevalidazione preliminare al deposito delle sentenze e sarà varato il *desk* del consigliere. È poi in corso di aggiudicazione la gara per la telematizzazione del processo penale, con un progetto esecutivo che potrebbe essere pronto già entro giugno 2019. Il corretto funzionamento della giustizia civile rappresenta uno dei capisaldi dell'ordinamento giuridico, giacché a esso è delegata la tutela dei diritti dei lavoratori, contraenti, imprenditori e creditori, nonché dei cittadini medesimi nelle loro vesti di genitori, figli e coniugi. Assoluto dovrà essere - lo è stato già in questi primi mesi - l'impegno del mio Dicastero per garantire un servizio in grado di produrre decisioni in tempi congrui e ragionevoli, evitando che l'accesso al processo civile si trasformi in una richiesta di giustizia costantemente negata,

l'obiettivo primario dell'attività del mio Ministero e del Governo è stato individuato in un intervento analitico, a carattere semplificatorio, sul processo civile. Al di là del *trend*, in aumento o in diminuzione, la statistica della giurisdizione civile ci pone di fronte a un dato obiettivo, ossia l'enorme richiesta di giustizia che proviene dai cittadini. Al 31 dicembre 2018 sono infatti complessivamente stimati in ben 3.215.989 i processi di nuova iscrizione in ogni grado di giudizio. Nonostante il notevole e meritorio sforzo posto in essere, giorno dopo giorno, dai magistrati, dal personale amministrativo, dagli avvocati e da tutti gli operatori del diritto e nonostante le numerose riforme che si sono succedute nel tempo, a questa domanda non è mai stata fornita adeguata risposta. Anzi - come ho sostenuto in altre sedi - la giustizia civile soffre di ipertrofia normativa. Le riforme sono state frettolose, episodiche e prive di un razionale coordinamento e hanno generato effetti più dannosi che favorevoli all'interno di una macchina estremamente complessa, richiedendo ulteriori tempi e sforzi giurisprudenziali per assorbire le modifiche e, paradossalmente, cagionando esse stesse ulteriori criticità e ritardi. Una riforma del processo civile deve dunque essere incentrata sui criteri della selettività, nonché della semplificazione normativa, provvedendo alla soluzione della complessità e delle frammentazioni che frequentemente rappresentano non garanzie per gli utenti, ma freni al corretto dipanarsi delle procedure. Entro la prima metà di febbraio 2019 sarà depositato un disegno di legge delega avente a oggetto la riforma del rito civile, unitamente alla riforma del rito penale. Per quanto riguarda la riforma del rito civile, il provvedimento introdurrà meccanismi semplificatori per le cause riservate alla decisione del tribunale in composizione monocratica e collegiale, per il giudizio dinanzi al giudice di pace e per le impugnazioni: insomma, un processo più semplice e comprensibile ai cittadini. Proprio la destrutturazione del processo rappresenta l'altra anima fondamentale del progetto di riforma, al fine di dar vita a una prima ipotesi di processo ispirato ai principi del *case management* nel quale sia consentito al giudice e alle parti di modulare tempi e adempimenti processuali sulla base dell'effettiva complessità della controversia e delle reali esigenze difensive, chiaramente nel rispetto dei diritti delle parti coinvolte nel contenzioso. Si tratterà di un processo che a me piace definire a fisarmonica, e cioè un processo che possa durare una o due udienze al massimo per cause semplici e che, invece, abbia un'estensione temporale maggiore rispetto a cause più complesse che richiedono, ovviamente, un approfondimento in sede di giudizio. Lungo questa direttiva l'intervento dovrà prevedere tra i criteri anche altri istituti in grado di comprimere i tempi del processo senza diminuire funzionalità e garanzie. Penso - ad esempio - all'obbligatorietà del deposito degli atti introduttivi con modalità esclusivamente telematiche. In tale ottica, anche l'istituto della mediazione obbligatoria sarà oggetto di un accorato *restyling* fondato sulla base della valutazione dei risultati che sono stati ottenuti nel tempo. L'altro grande ramo di intervento nella giustizia civile portato a compimento nell'anno 2018 è rappresentato dalla riforma sistematica delle procedure di insolvenza. Come è noto, l'11 ottobre 2017 è stata approvata la legge n. 155, contenente la delega al Governo per la riforma della disciplina della crisi di impresa e dell'insolvenza. L'adozione del decreto legislativo di attuazione della suddetta delega, il cui sistema è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri il 10 gennaio 2019, andrà a sostituire integralmente l'attuale legge fallimentare nonché la legge n. 3 del 2012. Anche in questo caso, l'approccio metodologico è stato basato sull'evidente necessità di rendere più rapida la risposta in materia fallimentare e meno farraginose le procedure, rese poco agili dal continuo sovrapporsi sovrapporsi di modifiche parziali e dalla conseguente difficoltà di armonizzare le disposizioni riformate e quelle rimaste invariate. La certezza dei tempi e delle risposte giuridiche rappresentano un volano per l'economia ed un fattore in grado di attirare capitali esteri. Ecco perché l'obiettivo dichiarato della riforma è stato quello di realizzare un moderno sistema dell'insolvenza

Sulla base di tale principio, si è deciso di sostituire il concetto di fallimento con quello di liquidazione giudiziaria. Il nuovo approccio lessicale, volto a evitare l'aura di stigmatizzazione sociale, anche personale, che storicamente il termine fallimento

nella convinzione che le condizioni di insolvenza e di crisi aziendale rappresentino momenti fisiologici dell'impresa, ma proprio per tali motivi prevedibili, sono state inserite misure di allerta che, permettendo di anticipare l'emersione della crisi, danno vita a una fase preventiva a una fase preventiva diretta a una rapida analisi delle cause del malessere economico e finanziario dell'imprenditore, destinata a risolversi, all'occorrenza, in un vero e proprio servizio di composizione assistita della crisi.

Quel progetto era stato sostenuto perché era nell'interesse dei cittadini e, coerentemente, una volta in maggioranza, abbiamo proseguito in quella attività, correggendo laddove era necessario, arrivando a un risultato importante per i cittadini. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Credo che questo rappresenti un esempio virtuoso, che riporta i cittadini a credere in una politica che non stravolga la loro vita e quella degli imprenditori a ogni cambio di Governo, ma prosegua, laddove possibile, e nei limiti della compatibilità con la nuova linea politica, su progetti realmente a loro favore. In piena sintonia con lo spirito riformatore, nell'anno 2018 l'attività ministeriale ha dato vita a ulteriori interventi normativi nel settore civile, attualmente *in* *itinere,* ispirati all'emergenza fortemente sentita di restituire snellezza a procedimenti burocratici quotidiani, favorendo il sempre minore accesso alle cancellerie o comunque agli uffici per gli adempimenti

una riduzione pari al 3 per cento sul totale dei procedimenti. Ora mi preme sottolineare - come ho già più volte detto - che il numero dei procedimenti è fondamentale, ma ogni volta dobbiamo chiederci cosa c'è dietro esso, consapevoli del fatto che, se la riduzione del numero dei contenziosi corrisponde a una rinuncia dei cittadini a richiedere giustizia, quello rappresenta il più grande fallimento dello Stato e nessun merito invece per il legislatore e per l'Amministrazione. *(Applausi dal Gruppo Per questi risultati sento il dovere di ringraziare pubblicamente la magistratura, il personale amministrativo, gli avvocati, i cancellieri e ogni altro operatore del diritto che hanno fornito un'adeguata risposta di giustizia a favore dei cittadini e dello Stato italiano. Quanto alla giustizia penale, essa ha rappresentato per anni il terreno di duri scontri politici, talvolta strumentali, i quali hanno impedito una serena valutazione delle criticità e delle priorità, producendo interventi di riforma poco incisivi e sporadici, di frequente dettati da situazioni emergenziali, facendo ricadere sui cittadini tutto il peso dell'inadeguatezza

Pertanto, in sintonia con le indicazioni già presenti nel contratto del Governo del cambiamento, l'intera azione ministeriale è stata incentrata sulle due fondamentali direttive della lotta alla corruzione e della riforma del sistema della prescrizione. Entrambi gli interventi normativi sono contenuti nella legge n. 3 del 9 gennaio 2019, la la cosiddetta spazza corrotti. I fenomeni corruttivi non solo rappresentano un grave ostacolo al tessuto economico sano del nostro Paese, limitando o scoraggiando gli investimenti, ma si pongono anche quale strumento che permette alle organizzazioni criminali, anche di matrice mafiosa, di avere un sostentamento e una maggiore attitudine alle alle infiltrazioni nel tessuto sociale, economico e politico dello Stato. Del resto, in materia di corruzione, i dati che provengono dalle statistiche internazionali sono allarmanti. Il livello di corruzione percepito nel settore pubblico è elevato e colloca l'Italia in posizione lontana dai vertici della classifica europea,

e sociali (Eurispes). Tale dato sfiora il 90 per cento e rischia di provocare conseguenze concrete sull'economia nazionale in termini di fiducia nelle istituzioni e nei mercati. Oltretutto, secondo la Banca mondiale, la corruzione costituisce uno dei maggiori ostacoli allo sviluppo economico e sociale degli Stati, incidendo negativamente sulla crescita, in misura stimata tra lo 0,5 e l'1 per cento annui. Nel dettaglio, nell'ultima graduatoria di Transparency International l'Italia figura al 69° posto, per cento degli italiani è convinto che istituzioni e politici abbiano a che fare con la corruzione. Questa non è un'opinione: questo è un dato oggettivo. E non è irrilevante il fatto che si tratti di una

Combattere questa vera e propria piaga sociale è allo stesso tempo un imperativo morale e un punto cruciale di un'azione politica che voglia proporsi di offrire ai cittadini l'immagine di una pubblica amministrazione efficiente e funzionale, nel pieno rispetto dell'articolo 97 della Costituzione. La riforma approvata presenta caratteri della organicità e della sistematicità, essendo stata pensata ed elaborata in modo da intervenire sul versante sia sostanziale che processuale investigativo, sul presupposto che una seria lotta alla corruzione richiede non solo un'adeguata strutturazione delle fattispecie incriminatrici, ma anche la scelta di strumenti di indagine

il cosiddetto Daspo per i corrotti e una speciale causa di non punibilità nel caso di volontaria, tempestiva e fattiva collaborazione. Parimenti sono stati forniti i nuovi strumenti investigativi agli organi inquirenti e all'autorità giudiziaria, attraverso l'estensione delle tecniche investigative speciali previste all'articolo 9 della legge n. 46 del 2006, segnatamente dell'agente sotto copertura, a una serie di reati contro la pubblica amministrazione, tra cui la concussione e la corruzione per l'esercizio della funzione, la corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, il traffico di influenze illecite. È stata altresì estesa alle indagini in materia di reati contro la pubblica amministrazione la possibilità della

di diritto sostanziale rimarrebbe effimero e meramente formale se, nonostante gli sforzi enormi degli operatori giuridici, non si riesce a garantire una risposta di giustizia in tempi certi e idonei a riaffermare il primato dello Stato. Nell'operare una sistematica riforma della prescrizione si è partiti dalle seguenti considerazioni di Il dato relativo al settore penale è davvero preoccupante ed evidenzia nel 2017 un tendenziale aumento dei processi che si estinguono per prescrizione: 9,4 per cento nel 2017 a fronte dell'8,7 per cento nel 2016. Nello specifico, i procedimenti prescritti sono sono stati 125.550, dei quali il 25,8 per cento in grado di appello. La ricerca della verità e l'esigenza di giustizia non possono essere frustrate dall'uso pretestuoso di un istituto che, pur avendo una funzione originaria nobile, non può però finire per assicurare l'impunità rispetto a comportamenti criminosi che provocano un elevato allarme sociale e, quando parlo di uso pretestuoso e strumentale, mi riferisco

sull'istituto della prescrizione, recuperandone e tutelandone l'autentica funzione di garante del diritto all'oblio del cittadino attraverso una modifica incisiva dell'articolo 159 del codice penale, introducendo una nuova protesi di sospensione del termine di prescrizione che si verifica al momento della pronuncia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna e prosegue sino alla data di esecutività della sentenza, che definisce il giudizio o irrevocabilità del decreto di condanna. In tal modo si è creato un punto di equilibrio tra esigenze di giustizia e quelle di chi legittimamente richiede di non essere soggetto di un procedimento penale per un tempo indeterminato. Si riafferma il principio per cui, a fronte di una sentenza di primo grado, lo Stato manifesta in maniera assoluta il suo interesse all'accertamento della verità. Allo stesso modo, si offre uno strumento di deterrenza rispetto alle strategie difensive meramente e legittimamente dilatorie in presenza di uno strumento fornito dalla legge. voglio rassicurare tutti coloro che sostengono che, allo stato dell'arte, la riduzione delle declaratorie assolutorie per prescrizione possa comportare un ulteriore allungamento dei processi. Vi garantisco che, proprio al fine di scongiurare tale rischio, è in programma sin d'ora un massiccio intervento sulle cause

in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, il cosiddetto codice rosso, che - mi preme dirlo - è stato scritto a quattro mani insieme al ministro Giulia Bongiorno. Tale iniziativa è volta a garantire l'assoluta tempestività degli interventi cautelari o di prevenzione a tutela delle vittime dei reati di maltrattamento, violenza sessuale, atti persecutori e lesioni aggravate, in quanto commessi in contesti familiari o nell'ambito di relazioni di convivenza, di pervenire, ove necessario, nel più breve tempo possibile, all'adozione di provvedimenti protettivi e di non avvicinamento e di impedire che possano ulteriormente porsi in pericolo la vita e l'incolumità fisica delle vittime di violenza domestica e di genere.

infatti, non dubito della compattezza delle istituzioni e delle forze politiche rispetto a una piaga sociale così grave. Passando al modello dell'esecuzione penale, tra la certezza della pena e la dignità della detenzione, oggi la situazione delle nostre carceri è drammatica. Ci sono stati già alcuni interventi che mirano a incidere su una situazione in cui i detenuti presenti negli istituti penitenziari al 21 gennaio 2019 sono 59.947, a fronte di una capienza regolamentare di 50.569

2018; gli eventi critici ammontano a 3.808 (473 ferimenti, 3.331 episodi di colluttazione, 2 tentati omicidi e 2 vere e proprie rivolte in carcere). Per garantire la razionalizzazione degli spazi e il miglioramento delle condizioni di vita dei detenuti in carcere, sono stati destinati cospicui fondi all'edilizia penitenziaria: ben 44 milioni di euro in più rispetto al passato, 85 milioni per il 2019 e 30 milioni per il 2020 quali residui presso il MIT del piano carceri precedente; per quanto riguarda il piano quindicennale, 80 milioni sono stati assegnati dal 2018 e 30 milioni è l'ammontare della nostra richiesta, nel quadro esigenziale, a

I fondi sopraindicati, tranne allo stato il residuo stanziamento relativo al piano carceri, possono essere investiti tramite le agevolazioni procedurali previste dal decreto-legge semplificazione all'articolo 7 che, nel dettaglio, per ovviare agli aspetti problematici connessi all'eccessiva lunghezza dei tempi intercorrenti tra la progettazione

flessibilità e ascolto. Mi preme sottolineare l'importanza che svolgono all'interno delle carceri i nostri agenti di polizia penitenziaria. *(Applausi che portano avanti non soltanto una funzione di sicurezza all'interno delle carceri, ma anche un'opera fondamentale di prevenzione per il tempo in cui i detenuti usciranno dalle carceri e dovranno essere reinseriti nella società. In questo senso l'attività che svolge la Polizia penitenziaria nel monitoraggio delle dinamiche che possono portare a incrementare fenomeni di terrorismo è fondamentale. È per questo che di recente abbiamo approvato la norma che prevede la possibilità per la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo di disporre direttamente di un *pool* di 20 agenti di polizia penitenziaria. Si tratta di un riconoscimento al loro lavoro e all'importanza del collegamento tra l'autorità giudiziaria, specializzata nella lotta alla mafia e al terrorismo, e gli agenti di polizia penitenziaria.

Il Governo si sta impegnando per cercare di incrementare le strutture che, a livello regionale, possano accogliere situazioni così particolari. Tra l'altro, ci siamo già attivati con il decreto sicurezza, approvando una norma

il perseguimento degli obiettivi prioritari dell'azione ministeriale in materia di lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, alla corruzione e al riciclaggio non può prescindere dalle azioni sul versante internazionale, ancor più in considerazione delle elevate aspettative riposte nella futura attività dell'istituenda procura europea. abbiamo assistito a una progressiva trasformazione delle realtà criminose, che hanno travalicato ormai ampiamente i confini nazionali. Oggi i principali fenomeni criminali e le attività illecite maggiormente lucrose e dannose per il tessuto economico sociale presentano una dimensione internazionale ed è pertanto richiesta una pari coesione di tutti i Paesi dell'eurozona dell'eurozona (e non solo) per dare vita a un'efficace azione di contrasto, approntando linee di intervento politiche e strumenti di lotta comuni e coordinati. Di conseguenza, per fronteggiare efficacemente l'aumento della criminalità transfrontaliera registratosi negli ultimi anni, questo Dicastero ha intensificato l'impegno nella cooperazione giudiziaria nel contesto dell'Unione europea, costituendo tra i punti cardine dell'azione ministeriale la lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata. Tra i più significativi risultati va menzionato il recente arresto del latitante Cesare Battisti, condannato in via definitiva alla pena dell'ergastolo. Egli è stato consegnato al nostro Paese dalle autorità boliviane, Paese dove si era rifugiato a seguito alla riforma del decreto di estradizione nei suoi confronti, siglato nel dicembre 2018 dalla Presidenza brasiliana, così fine alla lunga e complessa procedura attivata dalle nostre autorità e dal Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero che rappresento per assicurare il suo rientro in Italia. Fondamentale tappa raggiunta in questi mesi è stata l'adozione del regolamento istitutivo della nuova Procura

individuando i criteri di delega per la implementazione della direttiva UE 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, cosiddetta direttiva PIF (protezione interessi finanziari), e il regolamento EPPO. Entrambi gli schemi di disegno legislativo sono stati approvati dal Consiglio dei ministri in data 6 settembre 2018 e sono adesso al vaglio dell'*iter* parlamentare per verificare, su una materia così delicata, se devono essere apportate correzioni importanti. La procedura di nomina del procuratore europeo sta già costituendo

sono state viste come un significativo passo avanti del Paese nell'impegno nella lotta alla corruzione, nonché assolutamente adeguate a superare le contestazioni mosse dal Greco nel rapporto sul terzo ciclo di valutazione dell'Italia relativo alle incriminazioni e al finanziamento dei partiti.

Rispetto a tali iniziative - come sapete - il confronto con il Governo è stato assolutamente trasparente, franco e costruttivo.

addetti ai lavori. Un esempio di questo confronto auspico siano le riforme del processo civile e del processo penale. E, proprio in questo senso,

*(PD)*. Anche stamattina, come è naturale, giusto e doveroso, abbiamo ascoltato con estrema attenzione le comunicazioni che lei, signor Ministro, ha reso

Non parlo direttamente dei singoli temi, ma provo a partire - come ha fatto lei - in primo luogo da un metodo, da lei richiamato, peraltro giustamente, nella conclusione della sua ampia e lunga relazione. Lei ancora oggi ha lasciato intendere, ripetendolo più volte, che ascolto, confronto e collaborazione siano il suo metodo di lavoro, ma ancora oggi - esattamente come ha fatto tante volte negli ultimi mesi - per lei queste sono state parole vuote, prive di significato e di senso. Signor Ministro, lei ha detto che vorrebbe essere un Ministro che discute e ricerca il dialogo in Parlamento con le forze di opposizione, oltre che con la sua maggioranza, ma soprattutto un Ministro che ricerca il dialogo fuori, con i soggetti e il mondo della giustizia. Le faccio presente, però, che sicuramente sarà ricordato come il Ministro che a notte fonda ha portato in Parlamento, a insaputa dello stesso e senza dialogo e confronto con tutti i soggetti più autorevoli del mondo della giustizia, la riforma di un istituto molto importante nel mondo della giustizia, giustizia, la prescrizione. Lei è il Ministro che ha imbracciato il tema serissimo della lotta alla corruzione per usarlo esclusivamente come una medaglia politica da mettersi al petto anziché ascoltare - per esempio - le critiche, ma anche i validi suggerimenti che venivano dalla stessa autorità anticorruzione, oltre che dal suo presidente Raffaele Cantone. Lei è il Ministro che, di fronte a un Vice *Premier* che rivela di indagini ancora in corso per poi attaccare singoli magistrati che facevano il loro dovere, ha preferito tacere, anziché difendere l'indipendenza e l'autonomia della magistratura. Le chiedo: è questo sinceramente il modo con cui vorrebbe costruire le premesse del rispetto, del dialogo e della collaborazione reciproca con il Parlamento innanzitutto, con le forze di opposizione, ma anche con i principali soggetti operatori del mondo della giustizia? giustizia? Signor Ministro, ci dica per quanto ancora spaccerete a piene mani le buone intenzioni ispirate al dialogo se poi ogni evento e ogni provvedimento per voi è buono soltanto per diffondere rancore, sospetto e per costruire nemici da delegittimare? Lei crede veramente di fare un servizio alla giustizia italiana o di toglierla dal pantano politico - come spesso ha ripetuto - usando l'arresto di un crudele terrorista per mettere in piedi un'esibizione incredibile e indegna all'aeroporto di Roma, insieme al suo collega e *competitor* ministro Salvini? Questo per lei è il sistema della giustizia? Voi avete sporcato un arresto, che è il successo a lungo ricercato di tutte le Forze dell'ordine e di indagini italiane. Il vostro Governo dovrebbe imparare - mi consenta - la lezione di civiltà che vi hanno impartito il figlio di Torregiani e la poliziotta - lei vera, per fortuna - della Digos di Milano, che ha effettuato l'arresto di Battisti. Dato che questo è quello a cui ci avete abituato in questi mesi, oggi vorrei restare ai fatti. Nei primi mesi di questo Governo, molti sono stati i provvedimenti simbolo, fatti più che altro per rispondere alla volontà delle piazze, ma pochissimi sono stati quelli congegnati per portare effetti visibili e migliorare il nostro sistema giustizia. Prendo in considerazione quelli di cui voi andate più fieri. Lei ha detto - lo ha ripetuto anche stamattina qui in Aula - di aver risolto la senza misure straordinarie. Lei ha detto esattamente così, e lo ha ripetuto facendo riferimento alla mancata nomina di un commissario.

Oggi la situazione è che metà del palazzo di giustizia è stata trasferita in una sede che dovrebbe essere temporanea, ma da lei Ministro, non c'è notizia riguardo al nuovo polo sulla giustizia. Voglio ricordare che per il tribunale di Bari, penso che lei questo lo sappia, c'era un finanziamento consistente lasciato in eredità dal precedente Ministro della giustizia. Le chiedo: che fine hanno fatto quelle risorse? Sono ancora destinate a Bari oppure si sono semplicemente perse nei meandri dei milioni per l'edilizia giudiziaria che lei, Ministro, ogni tanto annuncia e poi dimentica di portare ad attuazione? Se lei vuole essere ricordato come il Ministro che passa dalle parole ai fatti, dia risposte concrete e predisponga finalmente un luogo idoneo ad ospitare, in via definitiva, il sistema della Giustizia penale barese. Fino ad ora sono stati troppi gli annunci a vuoto e molto, molto deludenti le iniziative reali. Lo dico perché anche nella legge di bilancio, da cui sarebbero dovuti arrivare - lei sostiene - stanziamenti epocali per il settore della giustizia, abbiamo visto soprattutto tagli consistenti ai programmi per l'amministrazione penitenziaria, per la giustizia civile e per la giustizia penale, tagli in controtendenza, a dir la verità, con gli anni precedenti. E allora, se vogliamo davvero parlare dell'aumento della pianta organica dei magistrati, diciamo pure - certo - che è e sarebbe un fatto estremamente positivo, purtroppo però solo se vi fossero, in corrispondenza, le necessarie coperture. Invece, e lei lo sa bene, in questa legge di bilancio si estende anche al comparto della giustizia il blocco delle assunzioni fino a novembre 2019. Ancora una volta, dunque, promesse vuote, promesse di facciata. Non prendiamoci in giro: voi state tagliando le risorse all'amministrazione della giustizia, promettendo qualcosa che in realtà state minando già da ora con le vostre scelte scellerate e irresponsabili. Ministro Bonafede, lei rischia di essere ricordato come il Ministro che, con la sospensione della prescrizione, ha dato un colpo definitivo al processo penale. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Nessuno ha ancora capito in che modo lo *stop* della prescrizione dovrebbe favorire la durata dei processi, né tantomeno lei ci consente di capirlo. Nessuno lo ha capito perché quella norma è un assegno scoperto sulle spalle degli italiani, che dal 2020 avranno processi infiniti e imputati colpevoli e comunque esposti alle pene a prescindere, perché la pena di un processo eterno è una pena a prescindere. Avreste potuto attendere i dati relativi all'intervento del 2017, come avrebbe fatto chiunque avesse a cuore davvero l'interesse della giustizia penale e non soltanto il proprio consenso. Questo Governo, invece, ha fatto uno scambio: abolizione della prescrizione in cambio di una riforma del processo di cui non si sa nulla, nulla! Questo rischia di chiudere in anticipo ogni spiraglio di confronto sul processo penale ma soprattutto rischia di chiudere la partita sulla depenalizzazione, faticosamente aperta negli anni precedenti, che richiede così di andare E invece scegliete la strada della criminalizzazione in chiave di consenso elettorale, così come siete andati dritti sulla prescrizione solo per mostrare un finto rigore, un pugno duro, senza però ascoltare la pioggia di critiche che proveniva da magistrati e avvocati, senza intervenire sostanzialmente sulla macchina e sul funzionamento della giustizia, su cui oggi ci saremmo aspettati, proprio per il tipo di relazione che lei doveva a quest'Aula e a questo Parlamento, parole più chiare, parole alle quali sarebbero dovuti seguire fatti. Lo avete fatto, per esempio, sull'anticorruzione, dove avreste potuto combinare, certo, repressione penale ma anche e soprattutto prevenzione, avreste potuto puntare, per esempio, su semplificazione organizzativa e trasparenza dei procedimenti amministrativi, perché è da qui che passa innanzitutto la legalità dei comportamenti, signor Ministro. E invece avete scelto la strada opposta, basata solo e soltanto sulla repressione dei fenomeni criminali, equiparando pericolosamente mafia e corruzione, come se fossero esattamente la stessa cosa. Peccato che mentre con una mano approvate l'anticorruzione, con l'altra consentite di derogare al codice degli appalti, alzando a 150.000 euro la soglia per l'affidamento diretto nei Comuni. I cittadini italiani devono sapere che questa è la vostra anticorruzione: con la mano destra utilizzate l'agente provocatore, utilizzate parole roboanti come DASPO e "spazzacorrotti" e con la sinistra fate norme apprezzatissime da tutti coloro che vorranno infiltrarsi illegalmente nelle amministrazioni locali. I risultati li vedremo. Ministro Bonafede, se guardiamo a come è stata amministrata la giustizia in questi mesi, io vedo certamente molte misure annunciate per il futuro, a cominciare da quelle sul processo penale civile e poche cose avviate, soprattutto nel percorso parlamentare. Vedo poi interventi simbolici

un percorso chiaro per raggiungerli. Questa è la mancanza più grave di questo Governo: avere contrabbandato palingenesi e finte rivoluzioni in cambio del nulla. Avete sacrificato sull'altare della propaganda e del consenso una civiltà giuridica tra le più invidiate d'Europa. Per questo le sue parole, oggi, confermano purtroppo la volontà di continuare su questa strada e per questo noi, come PD, vi diciamo: fermatevi. Fermatevi prima che sia troppo tardi. Proseguire così non è un dispetto che fate al Partito Democratico, non è un punto guadagnato a discapito di un avversario

colleghi, signor Ministro, ho ascoltato con grande attenzione la sua relazione e dalle sue parole risulta evidente come, seppur con minimi e impercettibili miglioramenti, restino pressoché inalterati i problemi endemici del sistema giustizia del nostro Paese: la lentezza dei tempi, l'efficienza e la produttività, nonostante l'impegno encomiabile di tutti gli operatori, cui va il mio e il nostro ringraziamento. I cittadini italiani avvertono come la giustizia sia ancora inadeguata e incapace di assicurare una tutela effettiva alla lesione dei loro diritti e dei loro interessi, con gravi conseguenze di sfiducia nei confronti dello Stato nel suo complesso. C'è un problema di risorse economiche per il funzionamento della macchina giudiziaria: l'Italia spende circa 90 euro per abitante, mentre la Germania ne C'è un problema di risorse umane: l'Italia ha circa dieci magistrati ogni 100.000 abitanti, mentre la Germania ne ha ben 23. Il nostro Paese risulta uno degli ultimi fra quelli appartenenti all'OCSE per lentezza delle cause civili. L'OCSE ha certificato che in Italia il tempo medio per la conclusione dei tre gradi di giudizio è pari a quasi otto anni, mentre la media degli altri Stati si colloca intorno a poco più di due anni. Il numero dei processi pendenti sia nel settore civile che in quello penale (rispettivamente più di tre milioni e mezzo nel civile e un milione e mezzo nel penale, secondo il monitoraggio del Ministero della giustizia), unito all'efficienza della macchina giudiziaria, determina l'impossibilità che questi siano definiti in tempi ragionevoli, così come stabilito dal secondo comma dell'articolo 111 della Costituzione. Le conseguenze sono un grave danno alla legalità, una generalizzata sfiducia nelle istituzioni e importanti ripercussioni economiche. Non solo. In Italia vi è un grande problema di credibilità del sistema giustizia, perché una sentenza penale che interviene dopo molti anni, che sia di condanna o di assoluzione, trova certamente le parti, sia il reo che la vittima, persone assolutamente diverse rispetto al momento della commissione dei fatti. Allo stesso modo, una sentenza civile pronunciata dopo tantissimo tempo produce effetti certamente attenuati fra le parti, se non fra i loro eredi addirittura. Su quali fronti occorrerebbe impegnarsi è noto. In tema di processo civile occorre ridurre al massimo i tempi dell'istruttoria per arrivare il più rapidamente possibile alla sentenza. In materia penale il problema della durata dei processi è ancora più grave, visto che da un lato apre le porte alla prescrizione dei procedimenti e dall'altro rischia di incatenare vittime e imputati, colpevoli e innocenti, a processi senza fine. Io non mi stancherò mai di ripetere che occorrono sentenze emesse nel più breve tempo possibile e una certezza dell'effetto risarcitorio della condanna, riaffermando la funzione rieducativa della pena e rafforzando le misure alternative. In questa occasione voglio riportare la sua attenzione anche su un tema che poco spazio ha nel dibattito del nostro Paese. La situazione delle carceri italiane versa in profonda crisi: a fronte di una capienza regolamentare pari a 50.632 detenuti, risulta un numero di quasi 60.000 detenuti, di cui almeno 10.000 in attesa di sentenza definitiva. L'Italia investe troppo poco, e da anni, sul funzionamento della macchina giudiziaria. Ci sono alcune misure particolarmente urgenti: ritengo che sia indispensabile procedere al completamento dell'informatizzazione dei processi in ogni ambito e settore e che bisogna fare in modo che lo sviluppo della macchina giudiziaria proceda di pari passo con l'innovazione tecnologica. È assurdo che in Italia non si possa avere un certificato di carichi pendenti che sia valido su tutto il territorio nazionale: l'unificazione dei carichi pendenti è qualcosa che si richiede da vent'anni e ancora non si è riusciti realizzare. Le notifiche via posta elettronica certificata, già proposte a questo Governo, sarebbero una prima soluzione per ridurre la lungaggine del sistema di notifica anche nel processo penale,

ancora ancorato a procedure obsolete. Ulteriori benefici, sia nei tempi che nei costi, potrebbero venire

telematiche, visto che molti rinvii di udienza sono determinati proprio dalla loro impossibilità a raggiungere i tribunali nelle date stabilite. Sono ancora molti gli ostacoli che si incontrano nel procedimento e che, senza aumentare le garanzie, producono un rallentamento oggettivo dei tempi del processo penale. Ad esempio, la disciplina del deposito degli atti alla fine delle indagini, con le notifiche, a volte a centinaia di imputati, e con la possibilità

che andrebbe quantomeno rivisto e circoscritto. Ho visto verbalizzanti che, dopo anni, sono stati costretti a ripercorrere tutte le fasi delle indagini, senza poter semplicemente confermare le complesse informative già rese in istruttoria, salvo naturalmente richiesta di ulteriori approfondimenti da parte degli operatori della giustizia. Non dimentichiamo che attualmente costruiamo due processi: un processo con gli atti garantiti, nell'istruttoria e nell'indagine, nel caso in cui l'imputato voglia ricorrere ai riti abbreviati o al rito immediato. Se però non si percorre quella strada, signor Ministro, che si va al dibattimento, si annulla tutto e si deve rifare tutto da capo. Sarebbe allora necessaria una scelta strutturale quanto epocale: o un processo inquisitorio garantito o un processo tutto basato sull'oralità, prendendo però tutto l'impianto del processo anglosassone, senza creare qualcosa che prende l'uno e l'altro modello e che naturalmente allunga i tempi del processo. Sarebbe infine necessaria, una volta per tutte, una revisione delle impugnazioni, non solo a livello di secondo grado, ma anche a livello di Cassazione. Concludo con un tema che mi è particolarmente caro: negli ultimi decenni sono stati inferti colpi notevolissimi alle organizzazioni mafiose, ma poiché la criminalità organizzata - come ha detto lei stesso, signor Ministro - mostra doti eccezionali di duttilità, di capacità di adeguamento ai tempi e di sfruttamento di nuove opportunità, l'evoluzione del metodo mafioso tra intimidazione, corruzione ed area grigia deve essere attentamente seguita, per prevenirne gli effetti. anche sul piano della cooperazione giudiziaria internazionale, che vede ancora non portate ad attuazione alcune Convenzioni sulla criminalità organizzata, come quella del 2000, che addirittura fu firmata a

un'attività proficua svolta da magistrati eccellenti, che ancora sono ricordati in tutto il mondo. La prevenzione consapevole, il monitoraggio, l'adeguamento della legislazione antimafia diventano quindi irrinunciabili e strategici. La lotta alle mafie non deve restare uno *slogan* per le campagne elettorali, deve essere una priorità per il Governo e il Parlamento.

abbiamo ascoltato con attenzione la sua relazione, che sicuramente era corposa e che immagino lei abbia un po' tagliato, rispetto a quello che era tutto il complesso delle pagine. Io non voglio utilizzare il mio intervento per ribadire quello che molti probabilmente ribadiranno oggi, cioè la questione del cosiddetto spazzacorrotti, che noi chiamiamo spazzagiustizia, e la questione della prescrizione. concentrare l'attenzione dell'Aula e naturalmente del Ministro, che ha svolto la relazione, su alcune questioni che seguono quel provvedimento e che si collegano poi alle prospettive che pare darsi questo Ministero.

il Ministro e il Governo ritengono di poter fare le assunzioni necessarie per far funzionare la macchina della giustizia.

Il cuore del problema sono le assunzioni detto che tutto può funzionare nel momento in cui le piante organiche previste per i magistrati vengono colmate e quindi si parte con la politica delle assunzioni. Ministro, noi abbiamo dei dubbi di carattere numerico che sono seri e che rischiano di inficiare tutto il disegno che lei porta all'attenzione dell'Assemblea e soprattutto del Paese,

Perché ho fatto questo ragionamento? Non per buttarmi in un ragionamento matematico, che non è mai stato la mia passione o la mia forza, ma per dire che il programma che lei ha in testa, rispetto alle riforme che si devono fare, non ha alcuna possibilità di andare in porto e rischia anzi di creare dei danni, per il semplice motivo che questi organici non sono riempiti sulla base di quello che noi leggiamo nella legge di bilancio. Si tratta di una questione sostanziale, dal momento che la giustizia non funziona perché non ci sono abbastanza magistrati, cancellieri e assistenti.

Quello che sarebbe dovuto essere l'atto più importante della legislatura o comunque dei primi sei mesi di Governo,

possa dormire tranquillo la notte, dopo aver presentato e fatto approvare una norma come quella che chiama spazzacorrotti, perché io, francamente, qualche problema di coscienza sulla prescrizione e su quello che avete fatto, me lo porrei tutte le sere.

devo dirle che, dopo averla sentita l'11 luglio in Commissione e questa mattina, mi verrebbe da complimentarmi con lei, perché lei ha la capacità di parlare e di illustrare dati,

Le dico subito, dunque, che mi vorrei complimentare perché lei è bravo a dire queste cose, ma poi non è conseguente nel dare le informazioni su quanto si vuole effettivamente fare. che l'11 luglio scorso, in Commissione, lei disse che l'azione del Governo del cambiamento, alla luce del contratto di Governo, si sarebbe svolta nel senso di dare una grande spinta all'amministrazione della giustizia, avendo individuato quali fossero le carenze della giustizia,

importante, cui lei ha fatto un piccolo accenno, è la magistratura onoraria. Ritengo che per la magistratura onoraria si debba trovare una perfetta soluzione, come peraltro voi auspicavate nel vostro contratto di Governo.

intervengo solo per dare contributi, non per criticare il Governo. Avremmo tante cose da dire. Lei ha parlato della giustizia di prossimità: pensa veramente che aprire degli sportelli in qualche Comune o in qualche decina di Comuni risolva il problema della giustizia di prossimità, quando lei sa benissimo, perché conosce il problema, che con la riforma della geografia giudiziaria importanti tribunali di frontiera sono stati soppressi e in quei luoghi non si può più rendere giustizia, sia per la situazione orografica in cui si trovano, sia per le distanze con il Comune capoluogo? Altro che che diano informazioni al cittadino! Abbiamo bisogno che la geografia giudiziaria venga rivista per dare la giustizia ai cittadini, perché oggi, come lei ha detto benissimo nella sua introduzione, in Italia vi è crisi assoluta e sfiducia nei confronti

che fare propaganda sulle azioni di Governo sia più utile che fare il Ministro della giustizia che risolve i problemi della giustizia. Mi riferisco alla riforma della prescrizione, che mi rendo conto attira di più: dire che con la sospensione della prescrizione si colpiscono i reati e i corrotti rende popolari, andiamo però a valutare attentamente

di esaurire un procedimento penale in venti anni, ma di quale giustizia parliamo? Se non strutturiamo bene l'amministrazione della giustizia e, addirittura, diamo la possibilità,

che riducono i tempi della giustizia, penso che faremmo un favore alla collettività. Lei ha poi parlato pochissimo di carceri.

Le diamo la possibilità, nella sua replica, di dirci qualcosa sull'edilizia carceraria, che ritengo sia un fattore importante non soltanto

Italia. Fratelli d'Italia presenterà una risoluzione, che stiamo preparando, in cui chiediamo degli impegni al Governo, sulle carceri, sulla prescrizione, sugli assistenti giudiziari,

Signor Presidente, colleghi, in quest'Aula così distratta mi rifaccio alle parole del collega Stancanelli, il quale ha detto che nella relazione del Ministro poco è stato dedicato alle questioni relative al carcere utilizzerò tutti i miei minuti solo per parlare di carcere. Nel corso del 2018, in coincidenza con i primi mesi del suo mandato, il Governo si è mosso, in materia di giustizia, in direzione diametralmente opposta rispetto ai Governi della precedente legislatura,

e neutralizzando quelle ancora in stato di completamento, ostacolandone o addirittura vanificandone la piene attuazione; in alcuni casi, come ad esempio quello dell'attuazione della delega in tema di riforma dell'ordinamento penitenziario, il Governo ha provveduto a superare lo schema già predisposto dal precedente Governo - e da questo già trasmesso alle Camere per il prescritto parere: eravamo appena insediati nel nuovo Parlamento e in Commissione giustizia, come primo atto, affrontammo questo parere. Il vostro Governo, signor Ministro, ha adottato un nuovo testo e ha eliminato le più significative innovazioni, determinando un grave arretramento sul tema delle garanzie dei diritti dei detenuti, ponendo nel nulla i punti di approdo cui si era giunti durante un evento importantissimo, che ha avuto un'eco e una risonanza non solo nazionale, cioè gli Stati generali dell'esecuzione penale,

Avete demolito il concetto di giustizia riparativa e lo avete fatto con furore ideologico, ritenendolo erroneamente a favore del reo e non invece a favore dell'offeso del reato, di colui che attende una risposta, una giustizia e una riparazione. Purtroppo è così, lo dovete ammettere: ciò che vi guida è il furore ideologico. Sì, un furore ideologico che ha travolto ed avvilito il principio, ma anche il precetto costituzionale della funzione rieducativa della pena. Onorevole Ministro, vorrei farle notare che quando il Ministro dell'interno, o meglio (come a me viene più spesso facile definirlo) il Ministro dell'inferno, ha dichiarato che un cittadino condannato per reati gravissimi deve marcire

Purtroppo, signor Ministro, non ho sentito alcuna sua replica a quella frase grave, offensiva e lesiva della Costituzione. Purtroppo ho assistito al suo teatrino: anche lei ha cominciato con il carnevale delle giacche e delle giacchette e, purtroppo, anche con l'uso anche con l'uso violento della lingua. Lei utilizza infatti l'espressione spazzacorrotti, ma le ricordo che anche i rifiuti si spazzano e che anche un condannato per corruzione è comunque un cittadino a cui la Costituzione riconosce diritti. Detto ciò,

che, lungi dall'assicurare maggiore efficienza al sistema di amministrazione della giustizia, invertono la tendenza positiva energicamente avviata nella scorsa legislatura, con una decurtazione che interessa principalmente i programmi per l'amministrazione penitenziaria e quello riguardante la giustizia civile e penale; per quanto riguarda, in particolare, l'amministrazione penitenziaria il Governo ha sostanzialmente vanificato la portata della delega sulla riforma dell'ordinamento penitenziario, e con la legge di bilancio assestato un altro fondamentale colpo alla ricerca di soluzioni normative che possano meglio adeguare il sistema alla finalità rieducativa della pena e in particolare, alla individuazione del trattamento, secondo la linea indicata dall'articolo 27 della Costituzione; in particolare, gli interventi restrittivi in tema di misure alternative alla detenzione dispiegheranno effetti perversi sulla condizione delle detenute e dei detenuti in condizione di particolare vulnerabilità, con specifico riferimento alle detenute madri e ai loro figli; Colleghi, di recente una delegazione di questo Senato si è recata a Rebibbia. A tale proposito, signor Ministro, mi rifaccio allo stanziamento del bilancio:

i bambini presenti nelle nostre carceri in compagnia delle loro madri: purtroppo, nessuno può tenerli fuori dal carcere, perché

Siamo tornati ai dati tristissimi degli anni del sovraffollamento, quando questo era più alto: vi ricordo che 66 suicidi accaddero nel 2010. Di tutto questo, che riguarda non solo la giustizia, ma soprattutto i diritti umani, nessuno s'interessa in questo Senato. Il precedente Governo aveva emanato una direttiva sulla prevenzione dei suicidi e i numeri erano calati: le chiedo ora cosa state facendo su questo, signor Ministro. Il mio pensiero va a tutti coloro che si trovano nelle mani dello Stato, perché quando un cittadino si trova nelle mani dello Stato, quest'ultimo è il garante della sua incolumità: non voglio ricordare Cucchi, Aldovrandi e i fatti recenti di Empoli. Anche i detenuti sono nelle mani dello Stato, che deve garantire la loro incolumità. Si deve Si deve quindi affrontare la situazione d'emergenza nelle carceri non solo intervenendo con un piano di edilizia carceraria. Non basta, non è sufficiente - lo dico anche al collega Stancanelli ma si deve intervenire sull'esecuzione della pena e sulle misure alternative alla detenzione, garantite non solo dalla Polizia penitenziaria - cui va il nostro ringraziamento - ma anche da tutti gli altri operatori della fase rieducativa e dell'esecuzione esterna. Le ricordo un altro fatto gravissimo,

il carcere, uomini e donne che hanno le competenze per farlo. Era dal 1969 (lei era bambino come me) che non accadeva un fatto del genere e su questo la sua voce non è giunta.

sui concetti di partecipazione e condivisione vogliamo lavorare per concretizzare quei percorsi che ha richiamato lei stesso e che - come ha giustamente evocato - devono avere una sola stella polare, la giustizia; non come semplice concetto, non come un feticcio, ma come un diritto dei cittadini a vedersi tutelati. Lei ha correttamente ricordato un aspetto molto triste: oggi il sistema giustizia genera nei cittadini un istintivo senso di sfiducia. Questo però non deve rimanere un cartellino da mettere sulla porta del tribunale. Faccio l'avvocato anch'io, sono civilista e tutti i giorni frequento le aule di tribunale e mi devo confrontare con i miei clienti che hanno problematiche quotidiane molto semplici. Non vado a parlare di grandi questioni, ma della vera giustizia, quella piccola giustizia che tutti i cittadini devono riuscire ad avere ogni singolo giorno. Sappiamo tutti che il personale della magistratura e dell'avvocatura ha delle eccellenze, come giustamente ha richiamato, ma mi permetto di fare un richiamo: se un campione di Formula 1 ha una macchina che non va, di certo non vince. Ecco allora che gli interventi che ha evocato per l'innovazione e l'organizzazione sono fondamentali, perché anni di *spending review* non hanno risolto i problemi in modo complessivo. Ben venga la razionalizzazione, ma stiamo attenti a non razionalizzare la certezza del diritto, che deve rimanere un baluardo della nostra civiltà giuridica.

a suo tempo la sezione distaccata di Desio, ma anche su Cuneo e su tantissime altre realtà la chiusura ha portato notevoli disagi nello svolgimento quotidiano dell'attività processuale. Ciò veniva fatto senza una vera e propria razionalità, ma semplicemente sulla base di un calcolo economico. Questo deve essere un monito importante, proprio perché bisogna salvaguardare quei presidi di legalità che giustamente lei ha ricordato. Sul punto degli uffici di prossimità, ho apprezzato il suo richiamo: presso il mio foro c'è già qualcosa di simile per quanto riguarda la volontaria giurisdizione e l'assistenza a tutte quelle persone che non hanno la possibilità di rivolgersi

che tutti i cittadini devono poter toccare con mano, e non necessariamente perché ci deve essere un problema grande; magari il problema è piccolo. Un cliente viene da me perché magari ha bisogno di un'amministrazione di sostegno poiché ha la mamma o il papà in difficoltà,

Se non ho annotato male dalla sua relazione, oltre 3 milioni sono i processi di nuova iscrizione. Credo che potrebbero essere anche molti di più, se quel sentimento di sfiducia di cui parlavamo prima non ci fosse. È proprio per questo che una riforma del processo civile è fondamentale. È buona la direzione sulla semplificazione, sulla compressibilità del processo: è ottima. In tal senso, come mi è stato insegnato dal mio maestro, bisogna imparare dagli altri perché se gli altri fanno meglio le cose dobbiamo imparare da loro, senza copiare. Penso ad altri ordinamenti, magari anche quelli di matrice anglosassone, che della speditezza e della celerità hanno fatto un loro baluardo giuridico:

un breve cenno all'intervento della giustizia in materia di diritto di famiglia. Faccio diritto di famiglia anch'io: l'assistenza alle famiglie è un aspetto importante,

possa essere attuata sia nelle aule di tribunale che per strada.

Una relazione del Ministro della giustizia come la voleva il ministro Castelli era semplicemente una riflessione collettiva sul sistema giudiziario, sulle necessarie riforme e non un'elencazione di quanto il Ministro ritiene di aver fatto o di piccoli richiami alle varie leggi e alle varie proposte. Occorreva un equilibrio tra la relazione, le opposizioni

con ampi spazi per i singoli parlamentari, al di là dei dieci minuti regolamentari, per poter intavolare un vero confronto sulla giustizia.

a cui lei ha solo accennato. La diminuzione delle cause non è per caso dipeso dall'aumento del contributo unificato? Forse, determinate persone che non hanno la capacità economica di sopportare un giudizio civile si si rivolgono ad altri sistemi di giustizia nella sua Sicilia o nella mia Campania e in altre Regioni d'Italia, che sono sistemi di legittimazione di contropoteri criminali che sono in condizione di garantire giustizia quando la stessa non può essere

del fatto che le preclusioni esistenti nel processo civile, introdotte negli ultimi anni per cercare di ridurre l'arretrato, avessero impedito l'accertamento della realtà processuale e del diritto. Oggi abbiamo queste lamentele. Io vorrei capire se il nuovo rito semplificato dà la possibilità al cittadino che non ha i mezzi per rivolgersi a grandi studi professionali di poter avere un accertamento giudiziale basato sul confronto processuale tra le parti del processo o no. Vede, bisogna sempre ragionare in termini generali e non per singoli casi. Passando

della norma costituzionale che prevede la ragionevole durata del processo e le devo dire che sono convinto che la prescrizione non sia, come lei ha detto, un diritto all'oblio:

proposito dell'aumento dei magistrati di cui parla, la collega Modena le ha già fatto presente quanto risulta dalla legge di bilancio appena approvata e quanto risulta dai concorsi che si possono bandire. Signor Ministro, lei deve tenere conto, quando parla di corruzione percepita e fa riferimento all'Eurispes, che lei è il Ministro della giustizia: è venuto a fare una relazione al Parlamento o sta facendo ancora campagna elettorale? La corruzione percepita

Paese. Lei non può combattere la corruzione percepita, potrà combattere, attraverso riforme serie, la reale corruzione nel nostro Paese, che è un cancro e un cancro va estirpato conoscendolo

Mi scusi, come fa a non tenere conto degli effetti della corruzione? Lei può combattere la corruzione solo conoscendone gli effetti ed eliminandoli.

Parlando sempre di penale, lei ha fatto riferimento ai suicidi in carcere e alle violenze. Esisteva una norma che aveva una sua efficacia di deterrenza, ma il vecchio Governo di centrosinistra l'ha abolita.

che la valutazione discrezionale del magistrato non determina alcuna deterrenza. E giustamente lei oggi cita l'aumento di alcuni atti di violenza avvenuti nelle carceri. Ho detto alcuni, ma stiamo parlando di centinaia, migliaia,

episodi di violenza all'anno da parte dei detenuti, con fatti gravissimi. Pertanto, bisogna tentare di individuare un sistema.

bambini in carcere. Signor Ministro, non esiste una norma, un atto che possa giustificare la detenzione dei bambini nelle carceri. Noi abbiamo lanciato un'idea: mai più bambini in carcere, e l'avevamo realizzata. Lei sa meglio di me che c'è l'ICAM di Milano e ci sono altre realtà. Bisognava trovare altre soluzioni. Non basta dire:

Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, ringrazio il Ministro per la sua relazione che mi dà la possibilità di intervenire, con la sua stessa emozione, su un tema a me molto caro, quello della giustizia, che ha impegnato alcuni anni della mia giovinezza come studentessa di giurisprudenza e riempie ancora le mie giornate nello svolgimento della professione-missione di avvocato. Sì, perché ritengo che occuparsi di giustizia sia una vera e propria missione e come diceva il giudice Rosario Livatino: «La legge, pur nella sua oggettiva identità e nella sua autonoma finalizzazione, è fatta per l'uomo e non l'uomo per la legge, per cui la stessa interpretazione e la stessa applicazione della legge vanno operate col suo spirito e non in quei termini formali». Penso che gli operatori del diritto comprendano il senso di queste parole, ma il compito della politica sia di farle comprendere ai cittadini. E questo Governo del cambiamento, che ha già messo le basi di un nuovo modo di intendere il rapporto tra giustizia, politica e cittadini, sta lavorando proprio in questa direzione. La mia esposizione non verterà sui temi dei provvedimenti *in itinere*, sicuramente apprezzabili verranno vagliati consapevolmente nella loro applicazione reale. Mi permetto di ribadire altri punti, come gli stanziamenti di risorse appena approvati con la legge di bilancio; risorse economiche che, al di là della loro consistenza, testimoniano l'attenzione volta ad assicurare l'amministrazione e il funzionamento del sistema giudiziario e il supporto ai tribunali civili, penali e minorili. risorse importanti per portare a compimento i processi assunzionali del personale dell'amministrazione giudiziaria in atto, coprire i posti vacanti in magistratura, garantire adeguati livelli di formazione del personale per migliorare la qualità dell'azione giudiziaria e amministrativa; elevare il livello di qualità e funzionalità degli edifici e dei servizi, innalzando anche gli *standard* di sicurezza e garantire la piena accessibilità delle strutture giudiziarie e penitenziarie alle persone con disabilità; realizzare una rete di sportelli e uffici di prossimità, presidi di legalità, per agevolare l'accesso ai servizi della giustizia a tutti, tenendo conto delle aree più disagiate del territorio, penalizzate dalla lontananza delle sedi giudiziarie. Ancora, ricordo che in pochi mesi è stata approvata definitivamente la riforma dell'ordinamento penitenziario, con l'introduzione di disposizioni importanti per adeguare le condizioni di detenzione al pieno rispetto della dignità umana, permettendo il recupero sociale e un controllo effettivo dei percorsi di risocializzazione. Particolare riguardo si pone sull'assistenza sanitaria, non solo confermando l'operatività del Servizio sanitario nazionale negli istituti penitenziari, ma garantendo il principio non scontato della parità tra detenuti e soggetti liberi nella tutela del diritto fondamentale alla salute. Si interviene con determinazione nelle disposizioni in tema di vita penitenziaria e lavoro, con misure volte ad integrare i soggetti più vulnerabili, come le donne e gli stranieri. Per le donne si afferma il principio, anche questo non scontato, della parità di accesso alla formazione culturale e professionale e per gli stranieri si prevede l'insegnamento della lingua italiana e finalmente un primo approccio ai nostri principi costituzionali, nonché l'inserimento, tra il personale dell'amministrazione degli istituti penitenziari, dei mediatori culturali e degli interpreti. Si rafforza in modo decisivo il ruolo del lavoro negli istituti penitenziari,

con una nuova politica per la giustizia minorile e una nuova organizzazione dei servizi minorili delle comunità pubbliche e private, implementando l'istruzione, la formazione professionale e l'inserimento nel mondo del lavoro all'interno e all'esterno degli istituti di pena, potenziando percorsi di inclusione sociale e l'attuazione dei progetti europei. Si ampliano i presupposti per le misure alternative alla detenzione, prevedendo anche un più ampio accesso alle misure alternative di comunità. Altra misura importante, delineata nelle linee programmatiche del Ministero, è l'*input* dato al nuovo codice in ordine ai temi della crisi d'impresa e dell'insolvenza, per salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro al fallimento dell'azienda. Si sostituisce, non a caso, come già è stato detto, il termine «fallimento» con l'espressione «liquidazione giudiziale», come avviene negli altri Paesi europei, proprio per evitare quella fastidiosa forma di discredito sociale, anche personale, che da sempre si accompagna alla parola «fallito». Si armonizzano le procedure di gestione della crisi e dell'insolvenza del datore di lavoro, con forme di tutela dell'occupazione e del reddito dei lavoratori. Occorre non solo risanare l'impresa, ma anche soddisfare i creditori. Si privilegiano, nell'ottica della tutela e del recupero dell'impresa, strumenti e procedure alternative a quelli dell'esecuzione giudiziale. sicuramente oggi non possiamo dire di aver cambiato il mondo giuridico e giudiziario, ma credo che questi accenni a quanto già messo in campo dal nostro Governo e dal Ministero della giustizia siano i primi passi verso la giusta direzione, che tiene conto, prima e al di là di ogni misura e riforma, dell'uomo in quanto persona e non come condannato, recluso o fallito e riscopre i princìpi fondanti della nostra Costituzione. Pertanto, concludo sicura che l'opera politica che portiamo avanti nel campo della giustizia ha come unico obiettivo assicurare migliori condizioni umane per tutti, senza più il conflitto perenne tra governo degli uomini e governo delle leggi, perché la dignità umana non può sfuggire al diritto, ma è al suo interno e deve guidare il sistema giuridico. La parola chiave della nostra politica e soprattutto delle azioni del Ministero della giustizia, per portare quel cambio epocale di paradigma, riducendo gli eccessi e gli arbitri del potere, è proprio «dignità umana», che ognuno di noi è chiamato a ricordare di avere per se stesso, ma soprattutto per poter veramente rispettare l'altro.

Signor Presidente, prima di passare la parola per i singoli pareri al sottosegretario Ferraresi, mi sono voluto concentrare nella raccolta

da chi, come il senatore Grasso, segnalava la lentezza di processi ancora a un livello

che secondo me è importante avere sempre come stella polare in qualsiasi azione che svolgiamo all'interno delle istituzioni: mi riferisco al dovere e all'onore di dire sempre la verità. La verità io la devo non soltanto a voi, ma a tutti i cittadini italiani. E la verità è che la nostra giustizia è in condizioni drammatiche: se io dicessi qualcosa di differente, sarebbe una presa in giro. Se io oggi dicessi che in sette mesi di Governo ho trovato le soluzioni a tutti i problemi della giustizia, dovreste offendermi e mandarmi a quel paese, perché in quel momento vi avrei semplicemente preso in giro. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Però posso dire che, per la prima volta, questi problemi trovano un Governo che da una parte risponde dove può nell'immediato, di fronte alle urgenze e alle emergenze, e dall'altra parte pone le fondamenta per un

senatrice Valente mi diceva che su Bari io non avrei parlato di urgenze e di emergenze. In realtà il mio ragionamento era riferito al discorso della mancata nomina di un commissario,

però, non è stata affrontata con la cultura dell'emergenza, cioè con la solita nomina di un superuomo, il commissario, che mandato lì, in deroga a tutte le leggi, avrebbe dovuto risolvere la situazione. Abbiamo messo un punto a questo

agli unici due problemi su cui non ho potuto dare una risposta adesso, perché intendo darla nell'arco dei prossimi due mesi, vista l'istituzione di un tavolo molto importante di interlocuzione e confronto

riguarda la graduatoria degli idonei assistenti giudiziari: sono perfettamente consapevole che ci sono delle aspettative importanti. Agli interessati più volte che non voglio promettere nulla in termini di dati e dettagli. Ho già detto che ci sarà uno scorrimento della graduatoria, con tempi e modalità che mi riservo di comunicare anche nell'arco dei prossimi due mesi, in quanto la prima urgenza

un Governo che non dà le risposte e non ci dice quanto spende. L'ho già detto tantissime volte e lo ripeto: il complesso dei soldi che sono stati investiti nella giustizia è stimato in circa 500 milioni di euro. su cui anche la senatrice Modena ha sollevato alcune perplessità, sono sotto gli occhi di tutti. Infatti, provvederemo anzitutto alla copertura integrale dell'organico della magistratura ma convinti che la giustizia debba richiedere un impegno in più. Abbiamo previsto previsto che nel triennio ci siano 600 magistrati in più rispetto alla pianta organica (ossia, oltre alla saturazione della pianta organica, ci saranno 600 magistrati in più) 3.000 unità di personale amministrativo, oltre a tutte le altre assunzioni che ho già menzionato. Si è poi parlato della situazione delle carceri. In tale ambito, è prevista un'assunzione di 1.200 agenti di polizia penitenziaria soltanto nel 2019. Possiamo vedere le prospettive in maniera differente - qualcuno sarà d'accordo e qualcun altro no, ci mancherebbe - ma non si possono negare dati oggettivi. Non si può negare la verità. La verità è che l'ultima legge di bilancio ha rappresentato un passo verso una nuova cultura della giustizia: un nuovo modo di concepire la giustizia come priorità di un Governo nell'interesse dei cittadini. Ciò è non solo inequivocabile, ma anche concreto, oggettivo e inserito, con lettere e numeri, nella legge di bilancio. Ci tengo anche a sottolineare il riferimento, che più o meno da tutti è stato fatto, al dialogo, all'ascolto al confronto. Giustamente la senatrice Valente sottolineava la vicenda legislativa dell'emendamento sulla prescrizione. Non dubito del fatto che in questi primi mesi di Governo ci siano stati dei momenti in cui il Governo ha dovuto accelerare, ma eravamo di fronte ad urgenze: urgenze di fronte alle quali il Paese non aveva più tempo. Perché non c'è più tempo di fronte ad un 30 per cento di cittadini che hanno rinunciato negli ultimi due anni a chiedere giustizia perché non si fidano della giustizia. Questo è un dato fondamentale. Questo è il punto di partenza! Come ho detto, il mio auspicio è che, prima di tutto, il primo importante orizzonte di confronto sia rappresentato dalle riforme del processo civile e del processo penale, dove proprio lo strumento della legge delega darà la possibilità al Parlamento di esprimersi e di avere un confronto nell'ambito dei tempi richiesti. Dobbiamo, però, ammettere che nei primi sei mesi ci sono state urgenze di fronte alle quali il Paese non poteva più aspettare. Noi ci assumiamo la responsabilità di aver individuato le priorità che dovevano essere portate immediatamente all'attenzione del Parlamento, pur volendo sottolineare che, comunque, la legge anticorruzione (la cosiddetta spazzacorrotti) è stata approvata a seguito di tre letture in Parlamento.

L'ottica è quella di non stravolgere il diritto ma di intervenire laddove è evidente che vi sono lungaggini che i cittadini non comprendono più.

Su questo punto tengo a dire che l'impegno c'è già stato perché, come lei sa benissimo, nei mesi scorsi, dopo un mio intervento a Vienna, la Convenzione ha avuto, grazie all'impegno italiano, uno *step* di applicazione in più che permetterà di verificare meglio quali effettivamente sapranno adattarsi e ottemperare a questo strumento, che fu voluto da Falcone. Mi creda se le dico che non c'è mattina in cui, entrando al Ministero della giustizia e trovandomi di fronte alla targa dedicata a Giovanni Falcone, sopra le scale che portano

e concludo - alla legge anticorruzione e alla prescrizione, è stato detto tanto. La senatrice Cirinnà mi rimprovera in qualche modo per l'uso del termine «spazzacorrotti», che però io rivendico. All'estero la legge è stata ribattezzata

dal Gruppo M5S)*: ogni volta che vediamo una parte di Paese impoverirsi di imprese che scappano all'estero lì c'è spesso un fenomeno di corruzione che disincentiva gli investimenti. Ogni volta che parliamo di ragazzi che vanno all'estero perché non trovano più meritocrazia, lì parliamo di corruzione. Ogni volta che a causa di un terremoto crolla un ospedale o una scuola, spesso si scopre che dietro quel crollo non c'è soltanto

e mi dispiace per la senatrice Cirinnà, per le domande che aveva fatto sull'edilizia penitenziaria, su cui avrei avuto piacere di rispondere. La senatrice Modena - mi pare - mi chiedeva se dormo la notte pensando all'anticorruzione.

il Paese ad un concetto di legalità che lo veda in una posizione di *leadership* a livello internazionale, perché la nostra magistratura, la nostra lotta alla corruzione, al terrorismo e alla criminalità organizzata rappresenta un'eccellenza a livello internazionale. Di questo ne dobbiamo andare orgogliosi e con orgoglio dico che quando vado nelle sedi internazionali non manco mai di sottolineare che noi, come Paese, abbiamo deciso di fare tesoro di un passato drammatico. Da quel passato abbiamo tratto norme all'avanguardia e per questo andiamo orgogliosi di essere italiani e di poter essere *leader* a livello internazionale

punto 2) il parere è favorevole con la seguente riformulazione: «a garantire un potenziamento - quantitativo e qualitativo - delle strutture carcerarie sul territorio nazionale sia attraverso l'implementazione di quelle esistenti sia attraverso l'edificazione di nuove».

punto 11) il parere è favorevole con la seguente riformulazione: «a sostenere, per quanto di propria competenza, l'approvazione in via definitiva della legge sulla legittima difesa». Sui

signor Ministro, sul fatto che uno dei grandi problemi della giustizia italiana sia la durata dei processi. Il buon funzionamento della giustizia e i tempi con cui uno Stato emette una sentenza rappresentano elementi sostanziali della qualità della democrazia. Com'è già stato detto, l'Italia ha la metà dei giudici della Germania, le strutture sono inadeguate, come ci ricorda la vicenda del tribunale di Bari, e le carceri sono sovraffollate. pertanto gli investimenti per le strutture, per il rafforzamento del personale amministrativo e per le nuove assunzione di magistrati. Un'altra causa, come lei stesso ricorda, è legata alla natura stessa dei procedimenti: troppo grande è il ruolo giocato dai formalismi, dalle eccezioni e dai vizi di forma adoperati soprattutto nel processo penale come strumento di difesa. Questo formalismo, sganciato dalla sostanza, è uno dei problemi più gravi del sistema italiano. Mi fa piacere, allora, sentire che l'obiettivo è semplificare le procedure. In questo senso, ben venga la riforma del processo civile da lei proposta, con un rito snello e con il rafforzamento del ruolo del giudice. Concordo anche con l'idea di abolire gli atti di citazione per sostituirli con i ricorsi, a patto che i giudici siano obbligati a fissare le udienze entro un certo lasso di tempo. Alcuni dei suoi predecessori hanno provato a risolvere questi problemi con grandi riforme che però in alcuni casi hanno addirittura aggravato i problemi. Per questo avevo apprezzato le sue parole in sede di Commissione nel corso dell'illustrazione delle linee programmatiche del suo Dicastero, quando ha annunciato una politica dei piccoli passi, proprio per non fare questi errori e per non costringere il sistema giustizia a un ennesimo stravolgimento. Insomma, Ministro, una bella teoria, che però è molto diversa dalla pratica di questi mesi. Fino a questo momento non avete rafforzato il ruolo del giudice, ma avete prodotto norme che limitano il suo potere discrezionale e che si prefigurano come vere e proprie norme-sentenza. Il caso più vistoso è sulla legittima difesa con la modifica dell'articolo 52 del codice penale, ma lo stesso vale anche con il decreto sulla sicurezza, con il restringimento dei casi di protezione umanitaria per gli stranieri, perché, a vostro dire, i giudici l'avevano applicato troppo spesso. Un'altra vostra caratteristica fino a questo momento è stata la leggerezza con cui avete maneggiato fondamentali princìpi giuridici Con l'introduzione di una norma, quella sulla revoca della cittadinanza, violate un principio fondamentale

spinge i cittadini a commetterli. E lo avete fatto con la norma sulla non punibilità del corrotto che denuncia un caso di corruzione. I pentiti in Italia sono stati importantissimi per alcuni processi, ma è anche vero che il pentitismo è stato adoperato da alcuni per sviare le indagini e per far ricadere su altri proprie responsabilità, determinando situazioni di vera e propria persecuzione giudiziaria. Quindi, tutto mi sembra tranne che una politica della prudenza e dei piccoli passi. Mi sembra invece una politica frutto di una precisa ideologia, la stessa che porta nel decreto spazzacorrotti - già il nome dice tutto - a inserire norme sui partiti, quasi a voler insinuare una correlazione tra politica e corruzione. In nome di questa visione ideologica avete introdotto la sospensione della prescrizione, senza però prima un intervento per velocizzare i processi. In questo modo probabilmente si andrà a ledere ancor di più il principio della giusta durata del processo. Signor Ministro, durante la sua audizione in Commissione giustizia aveva usato tre parole a suo dire chiave: ascolto, confronto e collaborazione. Mi chiedo dove sono finite, quando i penalisti hanno protestato sulla prescrizione; quando voci autorevoli si sono alzate sulle criticità del decreto sicurezza e della legge sulla legittima difesa. E dove rimane il suo confronto costruttivo con l'opposizione, quando poi dice che la volontà del popolo passa attraverso i voti di fiducia? Qualche giorno fa abbiamo visto un suo video su Facebook in cui si esibiva un latitante come un trofeo dì caccia. È un video che dà l'idea di uno Stato più interessato alla vendetta che alla ricerca della giustizia. Purtroppo quel video non è un errore di comunicazione ma rispecchia il quadro dei provvedimenti di questi mesi: provvedimenti molto utili sul terreno della spettacolarizzazione e della propaganda, ma scarsamente efficaci sul terreno di una giustizia che cerca di dare risposte giuste e rapide ai cittadini e che garantisce la certezza della pena. È la declinazione giudiziaria del populismo. Una giustizia che non ci piace, perché guarda con sospetto ai cittadini, perché non crede nelle potenzialità riabilitative della pena, perché mal sopporta l'idea che a scrivere le sentenze siano i giudici e perché risponde non ai problemi ma ai bisogni emozionali di una certa opinione pubblica. Una giustizia che - temo - renderà ancora più gravi i problemi del nostro sistema.

I numeri con i quali ho descritto tali problemi manifestano, però, l'urgenza di dover intervenire immediatamente. Il sistema giudiziario, com'è noto, permea di sé la vita dello Stato prima ancora dei suoi cittadini. civili, sociali, economici guardano infatti alla giustizia come alla loro autentica forma di garanzia e, di converso, il funzionamento della macchina giudiziaria condiziona il modo di vivere i predetti rapporti e, laddove manca la certezza del diritto, una comunità non può certamente prosperare. Come si può infatti richiedere a un investitore di fare impresa in Italia quando ciò comporta costi enormi, spesso dovuti a procedure farraginose e incomprensibili? Come possiamo chiedere ai cittadini di credere nella giustizia e di rispettare le leggi quando non sono certi che farlo corrisponda a vedere tutelati i loro diritti? Dagli stessi dati da lei riferiti, signor Ministro, si riscontra la sfiducia nella giustizia. Il decremento delle iscrizioni dei procedimenti, soprattutto in tema di lavoro, di procedimenti prefallimentari e di recupero crediti, insomma la decrescita dei procedimenti pendenti non è un fatto positivo, come lei stesso ha accennato, ma è correlato alla riduzione della domanda di giustizia per quasi tutte le materie. Non è accettabile che i processi siano vissuti come un girone dantesco e che sia «e fammi causa!» l'arrogante minaccia sempre più frequente da parte dei debitori per opporsi alla rivendicazione dei diritti. Non è un mistero che il nostro Paese sia afflitto da questa malattia, e che non si possa continuare a proporre, come avete fatto recentemente con la riforma della prescrizione - solo per citare l'ultimo e più clamoroso caso - interventi normativi *spot*, che non producono effetti strutturali sull'intera architettura del sistema, che ha bisogno, appunto, di una riforma complessiva. Sono molti i fattori che concorrono a determinare questo stato di cose. Conoscere le ragioni dei problemi è un presupposto essenziale per poterli risolvere. Con le sue parole, signor Ministro, lei sembra ammettere che questo Governo non solo non sia capace di produrre soluzioni credibili, ma che sia carente anche sotto il profilo dell'analisi delle criticità. Tra le priorità, Ministro, vorrei ricordarle le questioni relative agli interventi in tema di edilizia penitenziaria e di lavoro dei detenuti, sia intramurario che esterno, unico modo - è stato accertato da parecchi studi - per ridurre la recidiva e il ritorno al delitto: quindi, quella funzione rieducativa della pena che è alla base della nostra Costituzione. Vorrei poi ricordarle, signor Ministro, la magistratura onoraria: non ho sentito nella sua relazione alcun accenno a questa componente ormai irrinunciabile dell'amministrazione della giustizia, che ormai possiamo definire un precariato nella magistratura, non solo per definizione ma anche per trattamento. Forse è venuto il momento di rivedere tutto il sistema. Signor Ministro, la invito poi a non trascurare

quella dei detenuti che vengono trattenuti senza titolo nelle strutture penitenziarie per mancanza dei posti necessari individuati dalla legge. Infine, il tema della libertà di stampa e, in particolare, le norme sulla diffamazione e le querele temerarie richiedono un urgente intervento legislativo, già avviato nella scorsa legislatura, che va ripreso nella presente. Il funzionamento del sistema giustizia non può e non deve essere sacrificato sull'altare delle beghe e dei veti incrociati tra Lega e MoVimento 5 Stelle, com'è amaramente successo con il disegno di legge spazzacorrotti. Sarebbe grave, anzi, gravissimo se i propositi roboanti con cui riempite quotidianamente le vostre dichiarazioni non si traducessero in riforme utili e ben scritte. Molto del futuro del nostro Paese passa dalla capacità delle istituzioni di restituire ai cittadini la piena fiducia nello Stato. Purtroppo dobbiamo prendere atto che non avete ancora questa prospettiva. Per questo il voto di Liberi e Uguali non può che essere contrario alla risoluzione presentata dalla maggioranza. Prendo atto, però, che sono state accolte nella quasi totalità le osservazioni che abbiamo offerto al Parlamento e al Governo attraverso la nostra proposta di risoluzione e, convinti che ci sia ancora

il Ministro in replica ha ribadito di ascrivere a merito del Governo la legge cosiddetta anticorruzione e ha giustificato l'inserimento della riforma della prescrizione definendola una delle urgenze principali alle quali il Ministro, il suo Governo e la maggioranza hanno ritenuto fosse necessario e indilazionabile Ebbene, signor Ministro, lei sa benissimo che gli effetti in tema di corruzione della riforma della prescrizione si cominceranno a vedere nel nostro ordinamento,

fino al 2035 comunque nessun reato di corruzione si sarebbe prescritto, alla faccia dell'urgenza! Forse sarebbe stato meglio concentrarsi su quello che lei pure ha definito uno dei suoi obiettivi e cioè assicurare finalmente al sistema giustizia gli organici, gli strumenti, le dotazioni e il personale necessario, anche perché, signor Ministro, lei sa benissimo cento dei procedimenti penali la riforma che avete fatto non ha alcun effetto. Lei stesso ha detto che soltanto il 25 per cento dei procedimenti penali si prescrivono in appello e che tutti gli altri si prescrivono in istruttoria o, tutt'al più, in primo grado e quindi

di condanna. Signor Ministro, lei sa meglio di me che il 50 per cento di tutte le prescrizioni si verificano in quattro uffici giudiziari: Roma, Napoli, Torino e Venezia. Anziché fare una norma assolutamente propagandistica che comincerà ad avere effetto dal 2035, forse sarebbe allora stato meglio concentrarsi su questi quattro uffici giudiziari,

come uno strumento per far fronte alle manovre dilatorie degli avvocati degli imputati. Ebbene, signor Ministro, quelle che lei definisce manovre dilatorie sono legittimi esercizi di diritti costituzionali. Questa è la differenza tra il suo modo di concepire la giustizia e il nostro. Come se lei non sapesse che tutte le volte in cui si chiede un rinvio, già oggi il codice di procedura penale prevede la sospensione della prescrizione. Ma lei stesso, evidentemente, non crede a quello che dice infatti dice (e sappiamo che non sarà così) che i tempi non verranno dilazionati all'infinito, che i processi non verranno rinviati *sine die*, soprattutto in appello, e che lei metterà in campo tutte le azioni utili e necessarie a far sì che le condanne pesantissime che oggi lo Stato italiano deve pagare per effetto della legge Pinto non si verifichino più. che bisogno c'era di riformare la prescrizione. Da qui al 2035 sarebbe stato sufficiente fare quello che lei ha detto essere nel programma del suo Governo. Ed è molto pericoloso il messaggio che lanciate perché avete detto di avere abolito la corruzione grazie anche alla riforma della prescrizione. Un messaggio sbagliato che l'opinione pubblica potrebbe percepire in modo assolutamente errato. Come è sbagliato, signor Ministro, avere introdotto l'agente sotto copertura anche per la lotta alla corruzione. Siamo d'accordo sull'agente sotto copertura. Il fatto è che questo non è tale. Quello che avete introdotto voi è un agente provocatore vero e proprio perché la legge prevede addirittura che egli possa commettere attività prodromiche o strumentali e persino che possa offrire danaro al pubblico ufficiale per mettere alla prova la sua onestà. Questo non significa indagare per scoprire reati, bensì provocare i reati e lei sa meglio di me che questa è una norma incostituzionale che alla fine otterrà l'effetto opposto

nei Paesi di origine. Ebbene, eliminiamo la norma per cui è necessario il consenso del condannato per essere trasferito. Togliamola e mandiamolo a casa sua. Questo libererebbe enormi risorse da poter destinare agli agenti di polizia penitenziaria che lavorano in condizioni assolutamente disagiate, personale eroico che si sacrifica ogni giorno per garantire la sicurezza dei cittadini, lasciati nel dimenticatoio. *(Applausi dal Gruppo FdI)*. Mandiamo a casa loro, dunque, i detenuti stranieri senza chiedere il loro consenso e investiamo quelle risorse per l'edilizia carceraria e per il personale penitenziario. Ancora: lei ha parlato, signor Ministro, di ipertrofia normativa per quanto riguarda la riforma del processo civile. Noi sappiamo

Ebbene, certamente il numero eccessivo di riforme nel processo civile ha influito su questa lentezza. E tuttavia, signor Ministro, come si può pensare che il problema si possa risolvere cambiando nome all'atto di citazione e facendolo diventare un ricorso?

aggiungere un altro rito, quello per il giudice monocratico, possa essere una soluzione? In conclusione, colleghi, noi apprezziamo che la maggioranza e che il Governo abbiano accolto molte delle nostre raccomandazioni. Tuttavia questo, per le ragioni che ho detto e per molte altre che potrei citare, non ci consente di votare a favore della proposta di risoluzione della maggioranza.

signori del Governo, onorevoli senatori, la relazione che oggi è stata svolta conferma, ove ce ne fosse bisogno, l'assoluta incapacità di gestire un settore delicato come quello della giustizia. Oggi ho sentito dire che c'è stato un dialogo trasversale e un ascolto di tutte le parti, ma debbo dire che, se così è, qualcosa ci è sfuggito o forse ci sono davvero problemi di udito.

di legittima difesa. Di fatto, quella legge è esattamente il contrario di quanto hanno detto tutti i soggetti auditi in Commissione. Se questo è il modo di ascoltare, evidentemente qualche problema c'è. Inoltre, è inutile dare cifre sterili e fare petizioni di principio dicendo: «noi stiamo assumendo», «noi stiamo facendo concorsi», «noi stiamo potenziando il settore della giustizia». Non è vero,

E ancora, la confusione emerge in maniera chiarissima quando, nella proposta di risoluzione n. 2 della maggioranza, si dice che viene approvata la relazione sull'amministrazione della giustizia presentata oggi,

e chi governa il sistema giustizia non si è accorto dello stato in cui versa il sistema medesimo. A me dà l'impressione - l'ho ripetuto molte volte - che il Ministero si stia muovendo in questi mesi di governo con un unico obiettivo (che è stato negato oggi da un collega che stimo e apprezzo), quello cioè che risponde a un'idea molto demagogica: distruggere quanto era stato fatto nella precedente legislatura. per sovvertire l'obiettivo di mettere l'Italia al passo con i tempi e le direttive europee, e anche per evitare quelle procedure di infrazione che erano state aperte (qualcuna chiusa proprio grazie all'azione del Governo precedente). Invece sono sicuro che, andando di questo passo, qualche cosa a breve ci verrà rovesciata addosso e dovremmo ovviamente affrontarla. Si pensi alla situazione delle carceri, che certamente non ha non ha prospettive molto buone. A ben vedere, l'azione che sta portando avanti il Ministero e questo Governo, che viene annunciata sempre con proclami e atteggiamenti trionfalistici,

sono motivi ideologici o forse davvero c'è una scarsissima conoscenza delle problematiche vere, che gravitano intorno al sistema della giustizia.

sono perennemente in sciopero contro i provvedimenti che vengono propinati in questa Assemblea, senza alcuna possibilità di dialogo e di confronto, perché abbiamo una maggioranza che rimane silente e accetta passivamente le regole e dal Gruppo PD)*, che non consente neanche di alzare minimamente la testa in Commissione. Sono infatti convinto che molti dei colleghi, a cui ribadisco apprezzamento e stima, sono persone preparate, ma non possono aprire bocca, perché il Governo glielo vieta: questa è la verità. verità. Qualche problema, allora, esiste nella gestione del sistema giudiziario. Voglio credere che il Ministro sia a conoscenza del malessere diffuso tra tutti gli operatori del settore giustizia.

che abbiamo creato noi, classe politica, e alla quale però la stessa classe politica deve finalmente porre rimedio. Non mi pare però che ci sia nessuna volontà, al di là delle petizioni di principio, da parte di nessuno nel Governo. Governo. Un altro classico segnale del modo davvero molto superficiale con cui si affrontano i problemi è quello relativo al tribunale di Bari. Ci fa piacere che il tribunale di Bari non debba più lavorare nelle tende e che sia finito in un appartamento. la giustizia non si amministra così. La giustizia ha necessità di tempi seri e veri e allora proviamo a partire immediatamente. Non basta trovare un buco in cui far andare a lavorare coloro che, con grandissimo sacrificio, reggono in piedi il sistema giudiziario. Troviamo una soluzione,

reggono questo sistema. il codice sotto il braccio, questo sistema si fermerà. Se questo non accade è grazie al buon senso di tutti gli operatori, ma aiutiamoli e utilizziamo i mezzi che abbiamo a disposizione. Non fermiamoci alle mere petizioni di principio. Non c'è stato solo il provvedimento abnorme sul tribunale di Bari, ma ce ne sono tanti altri, che stanno già producendo effetti catastrofici, che fanno il paio con l'azione di Governo in qualsiasi altro settore, che sta causando una retrocessione in tutti i campi: si pensi all'economia, al lavoro e alla sicurezza. Si pensi ad esempio al cosiddetto decreto sicurezza, che ha ristretto in maniera inopinata il diritto di difesa e ha irragionevolmente pregiudicato in maniera significativa la libertà personale dell'individuo. Si pensi a quello che la maggioranza ha pomposamente chiamato decreto spazza corrotti, con un inutile inasprimento delle pene per i reati contro la pubblica amministrazione e che ha ristretto ulteriormente le garanzie di difesa,

alla modifica della disciplina della prescrizione, che produrrà uno spropositato allungamento dei processi. Si tratta di provvedimenti demagogici, che dimostrano, ancora una volta, l'assoluta scarsa conoscenza dello stato reale del sistema giustizia in questo Paese. Ma, anche in questo caso, la maggioranza ha subìto questi provvedimenti in silenzio e senza possibilità alcuna di alzare la testa. Si "scodellano" provvedimenti preconfezionati, negando qualsiasi possibilità di dialogo, al di là della capacità di ascolto che è stata qui affermata. Un'ultima annotazione riguarda la legge di bilancio, che è stata approvata frettolosamente e senza neppure aver avuto la possibilità di leggerla. È grave che la maggioranza si sia piegata ad accettare una cosa di questo genere, salvo poi sentirci dire che si stanno stanziando risorse ingenti a favore del sistema giustizia. Non è vero. Stranamente, tutte le assunzioni sono state bloccate (ho già detto prima da chi erano state avviate quelle procedure di assunzione); abbiamo le assunzioni bloccate fino al novembre 2019 e una serie di problemi che rimangono irrisolti, come quello dell'edilizia giudiziaria e dell'edilizia penitenziaria. Sono irrisolti: al di là delle petizioni, non c'è nulla di concreto, perché ci vuole danaro, che questo Governo non sta mettendo a disposizione del sistema. sistema. Anzi, in molti casi si è avuta una seria decurtazione delle risorse. Il personale non basta: si pensi ad esempio a cosa cagionerà l'introduzione della cosiddetta quota

già vessato dalla cronica carenza di personale, ci ritroveremo ancora alla paralisi di molti uffici. Insomma, in tema di giustizia l'attività del Governo è evidentemente connotata dalla scarsissima conoscenza delle vere problematiche e, soprattutto, dall'incapacità di affrontarle e di risolverle. A questo punto, non mi resta che dichiarare il voto favorevole alla proposta di risoluzione presentata dal Partito Democratico. Democratico. Non sono in condizione di dire alcunché circa le altre proposte di risoluzione, perché non ho ben capito (c'è stato un attimo di confusione, che credo sia stato condiviso da tutti); quindi valuteremo una volta

ha mosso dentro di noi una consapevolezza: finalmente un Ministro della giustizia che ha il coraggio di dire come stanno realmente le cose. Di questo la ringraziamo. La logica conseguenza di questa sua considerazione - che purtroppo, ahimè, noi condividiamo - è che questa maggioranza di Governo ha una responsabilità estremamente importante in tema di giustizia. Quest'ultima risponde a esigenze primarie dei cittadini, ma direi degli esseri umani. Non serve scomodare Foscolo, con «nozze e tribunali ed are», per ricordarci che siamo il Paese culla del diritto (le 12 tavole hanno 2.500 anni); e, da culla del diritto, non vogliamo certamente diventarne la bara. allora che il Governo abbia intrapreso la strada corretta, quella di un mutamento di campo di natura antropologica. Veniamo da una stagione in cui le vittime venivano trattate da colpevoli e i colpevoli da vittime; veniamo da una stagione in cui si sono tentate riforme della giustizia di natura strombazzatamente epocale, che poi in realtà diventavano dei topolini normalmente a costo zero. Dobbiamo cominciare finalmente ad approcciare la giustizia con una corretta visione antropologica. Non possiamo più permetterci una giustizia che dà ragione a tutti e finisce così con il non dare più giustizia a nessuno. Non possiamo più permetterci una giustizia che deve servire agli avvocati, ai magistrati o agli operatori del diritto: la giustizia deve essere al servizio dei cittadini. Questo capovolgimento antropologico passa attraverso un sentimento molto chiaro che è proprio di tutti i nostri cittadini: dall'anziano truffato e scippato, al bambino malmenato all'asilo, alla ragazzina costretta a sposare un uomo molto più vecchio di lei, fino alla banalissima lite di condominio, che pure è capace di muovere nell'animo delle persone sofferenze anche molto profonde. condividiamo con lei la prospettiva e partiamo da un principio che, per quanto riguarda il diritto penale, così recita: certamente l'umanità è recupero verso chi sbaglia, ma chi sbaglia paga.

Offrire celerità di risposta deve essere esigenza primaria dell'azione di Governo e condividiamo con lei questa volontà, così come condividiamo la necessità della preparazione affinché la giustizia sia non solo rapida, ma anche efficiente e di grande qualità. Questo potrebbe passare, ad esempio, anche per la preparazione multidisciplinare, con una formazione congiunta tra l'avvocatura, la magistratura e gli altri operatori del diritto, in modo che si parli la stessa lingua

Devo dire che personalmente mi è molto piaciuto il richiamo alla solennità e all'autorevolezza dei luoghi dove la giustizia viene amministrata, perché per il cittadino vedere lo *iuris dicere* in un luogo confacente

voce. Per quanto riguarda il processo civile e la riforma cui lei ha accennato, vorrei darle la certezza che il Gruppo della Lega al Senato è pronta a collaborare con lei e a dare tutto il suo contributo perché la riforma sia il più possibile ampia condivisa e vada incontro alle esigenze dei nostri cittadini. Allo stesso modo, per quanto riguarda il processo penale siamo assolutamente convinti della necessità di trovare un contemperamento tra l'esigenza della certezza della pena e la ragionevole durata del processo, entrambi princìpi costituzionali inderogabili. Siamo altresì convinti della funzione anche espiativa della pena. Infatti, è vero che la pena ha una funzione rieducativa, ma ha mille altre funzioni, tra cui quella espiativa.

che Ministri della Repubblica si siano recati in aeroporto per mostrare la presenza dello Stato che, finalmente, dopo anni di prese in giro, è stato in grado di fare giustizia.

fondamentale della polizia penitenziaria, che dipende dal suo Ministero e alla quale va tutta la nostra gratitudine. *(Applausi quotidiano, oserei dire quasi missionario, che gli agenti di polizia penitenziaria si trovano a svolgere, adempiendo sia alla funzione che è loro propria, cioè quella della custodia

la responsabilità cui ho fatto cenno all'inizio è davvero una responsabilità importante che abbiamo. Lei ha parlato di interlocuzione costante con il Parlamento. Noi le crediamo, perché nella legislatura che ci ha preceduto lei è stato tra banchi e, come noi, aveva il desiderio di portare idee, intuizioni e proposte per migliorare davvero la vita dei nostri cittadini e per fare della giustizia italiana quel fiore all'occhiello che tutti noi vorremmo fosse. Ci consideri, allora, nel Parlamento, e particolarmente nel Gruppo del Senato, un

Per questo motivo abbiamo preso buona nota di alcuni punti principali e quello che più mi ha colpito, perché si è verificato sin dalla prima fase del suo intervento, è stato il fatto di

Un altro punto è che noi abbiamo condiviso alcuni propositi che lei ha manifestato ma poi osserviamo che, dal manifestare questi propositi al metterli in pratica, c'è stato o un blocco oppure, addirittura, si è andati in direzione opposta. Iniziamo dalla questione della rapidità della giustizia, sia penale che civile. Su quella penale lei ha addirittura manifestato un proposito ambiziosissimo. Ha detto che vuole azzerare il capitolo di spesa della rifusione dei danni attraverso la legge Pinto, che è quella che rifonde i danni alle persone che sono state danneggiate dalla irragionevole durata del processo: addirittura, li vuole azzerare. Poi, però, voi avete approvato la cancellazione della prescrizione, che va contro i princìpi della Costituzione e contro i princìpi internazionali visto che, già prima di questo provvedimento, siamo stati più volte condannati a livello internazionale per l'irragionevole durata dei nostri processi. Così però si dice una cosa

anziché arrivare a condanne in tempi ragionevoli. Basterebbe leggere Cesare Beccaria che scriveva duecentocinquanta anni fa; cerchiamo di aggiornarci almeno alla metà del XVIII secolo, non torniamo più indietro di quello. Ebbene quelle persone innocenti, che subiscono un processo e che non vedono mai arrivarne la fine, magari perché qualcuno appositamente non lo fa finire. Le leggi e i princìpi costituzionali sono fatti nel presupposto che non tutti siano perfetti

e io la ribadisco all'Assemblea nel rispetto maggiormente delle opposizioni; se si può abbassare il tono della voce, permettiamo al senatore Malan di concludere il suo intervento. *(Applausi dal Gruppo

se non addirittura di diritto - va esattamente nella direzione opposta. Vuol dire che degli innocenti vengono rovinati in nome del popolo italiano, perché purtroppo questo è quello che avviene;

forse vengono proclamati innocenti. Comunque, sempre ricordando Cesare Beccaria, anche per i colpevoli la punizione deve essere il più possibile vicina al momento della commissione del fatto, anche per evitare di punire persone che ormai sono diverse quando passa troppo tempo, e comunque non costituire alcun deterrente. la giustizia civile, cito il contratto di Governo che lei giustamente ha citato più volte. Nel contratto c'è una frase che è straordinaria: «occorre velocizzare e snellire il processo civile mediante una semplificazione e riduzione drastica del numero dei riti, limitandoli al rito ordinario e al rito del lavoro». si dice che bisogna fare processi più brevi, ma poi si escludono tutti i riti abbreviati, lasciando solo il rito ordinario. Lei ha parlato adesso di questo progetto che speriamo di vedere presto, che dovrebbe mettere in atto lo strano principio contenuto nel contratto di Governo, del processo della formula a fisarmonica. Attenzione che la fisarmonica è uno strumento molto difficile e faticoso da usare, se già adesso con gli strumenti ordinari, abbiamo quelle lungaggini spaventose, che rappresentano uno dei principali motivi di mancanza di competitività dell'Italia e, in altre parole, del fatto che i posti di lavoro si trasferiscono all'estero; anche se è vero che poi darete il reddito di cittadinanza avendo un decimo dei soldi necessari nel frattempo si perdono posti di lavoro e, senza il lavoro, non si produce non c'è il denaro per realizzare nessuna delle iniziative che si vorrebbero fare. La realtà della giustizia di oggi è fatta di tanti aspetti di cui non abbiamo sentito parlare.

un minore si evolve rapidamente e dopo un po' non è più minore. Ci sono minori affidati a istituti la cui efficacia è spesso dubbia, che vivono praticamente per tutti i loro primi diciotto anni in situazioni provvisorie, senza che vengano rispettate le procedure. E poi ci dite che forse valutate l'opportunità di occuparvi di quel problema. C'è poi il problema della geografia giudiziaria, che ha fatto bene ad affrontare. Vediamo di arrivare ai fatti perché ormai avete fatto otto mesi completi di Governo. Non è che governerete per cent'anni in questa legislatura. C'è chi parla di tempi lunghi, ma di solito non porta molto bene parlare di tempi lunghi. C'è il problema dell'edilizia giudiziaria e anche su questo servono i fatti: con tutte le leggi sul raddoppio, quadruplicazione e decuplicazione della pena, dovrete triplicare come minimo l'edilizia giudiziaria. Bisogna farlo perché è paradossale che ci siano detenuti in in carcere per avere violato la legge (a volte sono solo in carcere in attesa di processo) e che si trovano in carceri contro la legge, tant'è vero che poi lo Stato italiano viene condannato e devono pagare tutti i contribuenti per queste gravissime carenze. Ci sono tanti problemi che affrontano i cittadini; ad esempio è stata anche citata da un senatore della maggioranza la questione dell'amministratore di sostegno, una ottima legge approvata in quest'Aula con l'intento di semplificare tutto e invece, sua applicazione sbagliata ho anche presentato un'interrogazione) per avere un sostegno che dovrebbe essere rapidissimo, quasi automatico fatti salvi i dovuti accertamenti, si aspettano molti mesi, anni e a volte molti rinunciano. Anche in questo caso ci sono aziende che chiudono perché non si riesce ad avere un amministratore di un amministratore di sostegno per una persona che non è in grado di esercitare le sue funzioni. Questi sono i veri problemi; non sono quelli della giustizia spettacolo, di fare comunicazione. Per carità, fate comunicazione, siete molto bravi, ma bisognerebbe anche avere qualcosa di concreto da comunicare. ha parlato di confronto costruttivo con le opposizioni. Sul cosiddetto provvedimento spazza corrotti (in realtà spazza giustizia), sia le opposizioni sia la maggioranza in Senato non hanno potuto modificare nulla e questo è stato anche fatto capire poco fa in un intervento.

Sulla *class action* già sappiamo che non ci sarà alcuna possibilità di intervento in Senato, né da parte della di maggioranza né dell'opposizione; in generale non è mai stato approvato un emendamento di Forza Italia in Commissione giustizia

a un'azienda segnalata come in difficoltà? *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Nessuna banca, perché a sua volta il funzionario rischierà qualcosa. L'Agenzia delle entrate viene anche coinvolta, per cui se un poveretto è in ritardo con un pagamento dell'IVA, magari perché la pubblica amministrazione non gli paga i crediti che ha, questa persona viene segnalata, le banche gli chiudono tutti i fidi e tutte le linee bancarie e questi fallisce. Sono cose terribili, disastrose. Il punto è che la giustizia (e il governare in generale) è un lavoro molto difficile, molto più difficile che

Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio il Ministro per la puntuale relazione sull'amministrazione della giustizia. La legislatura è iniziata da pochi mesi ed è chiaro l'intento riformatore che il Dicastero ha impresso nella sua azione di Governo. Come è noto, il contratto del Governo del cambiamento lancia uno sguardo complessivo al sistema giustizia, con una prospettiva che abbraccia un periodo ampio, cadenzato da una serie di innovazioni e di riforme, la cui iniziativa è equamente suddivisa tra Esecutivo e Parlamento. L'azione del Ministero che lei, signor Ministro, rappresenta abbraccia tematiche di così ampio rilievo, sia a livello costituzionale che di tutela dell'individuo, sia come persona sia come soggetto inserito in una comunità, che non può essere valutata negativamente, come abbiamo sentito in quest'Aula, se non dopo il decorso di un lasso di tempio più ampio per verificarne l'azione. Fino ad ora il Ministero e la Commissione giustizia hanno esaminato e approvato in via definitiva provvedimenti fondamentali per il sistema giustizia. Inizierei con un plauso in relazione alle ultime novità inserite in legge di bilancio: bilancio: gli interventi proposti nel settore giustizia mirano nel complesso al miglioramento dell'efficienza dell'amministrazione giudiziaria e riguardano essenzialmente il personale, perseguendo l'obiettivo della copertura e dell'ampliamento delle piante organiche, nonché della riqualificazione del personale stesso in servizio. L'obiettivo è finalmente quello di raggiungere la funzionalità del comparto giustizia, ormai gravato da annose inefficienze divenute croniche e purtroppo endemiche. Viene prevista l'assunzione a tempo indeterminato per il triennio di un numero massimo di 3.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale, onde evitare una sostanziale paralisi del sistema giustizia. Chi opera nel settore sa quale carenza di organico i tribunali siano costretti a sopportare e conosce l'importanza rivestita dalla categoria dei soggetti che si intendono assumere. Ricordiamoci che purtroppo a rimetterci per le inefficienze del comparto è sempre e soltanto il cittadino. Inoltre, l'organico della magistratura ordinaria viene aumentato di 600 unità. Unitamente a ciò, il Ministero bandirà annualmente per il triennio un concorso annuale per un massimo di ulteriori 200 posti. Le assunzioni sono state predisposte anche per il settore della giustizia amministrativa, dell'Avvocatura dello Stato e della giustizia contabile, altri settori essenziali. A nostro modo di vedere, importante è l'autorizzazione di spesa, in relazione alla riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria. L'incremento dei fondi destinati alle vittime di reati violenti e di quello di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonché agli orfani dei crimini domestici rappresenta una vittoria per questo Parlamento. Ricordo ancora le difficoltà provenienti dall'attuazione delle deleghe scaturenti dalla legge n. 103 del 2017, assolutamente distoniche rispetto a un efficace trattamento rieducativo del condannato. Il lavoro istruttorio compiuto dalla Commissione giustizia in sinergia con il Ministero ha favorito un'elaborazione compiuta dei testi dei vari decreti legislativi, allineando il trattamento rieducativo del reo a una maggiore sicurezza sociale. Fondamentali, al fine di garantire efficienza al sistema, sono anche le assunzioni di personale di Polizia penitenziaria ed i futuri progetti di edilizia penitenziaria sia nell'ambito dei lavori di ristrutturazione straordinaria degli impianti esistenti sia nella costruzione di nuovi. Questo mira a riallineare il sistema penitenziario italiano alle molteplici pronunce in ambito CEDU (Corte europea dei diritti dell'uomo), che hanno inesorabilmente condannato il nostro Paese a risarcimenti cospicui nei confronti di condannati detenuti in esecuzione di pena in condizioni inumane e degradanti, a causa della mancanza di spazio vitale nei luoghi in cui sono ristretti. In bilancio sono stati stanziati fondi per riuscire a implementare finalmente riforme organiche dei sistemi processuali, senza tralasciare il lavoro portato avanti sulla giustizia minorile. Con l'entrata in vigore dell'ordinamento penitenziario minorile viene rafforzato l'assetto delle misure alternative alla detenzione. Ne derivano sia notevoli vantaggi sul piano del contenimento della recidiva sia un abbattimento dei maggiori costi derivanti dagli oneri connessi alla gestione dei detenuti. La riforma del processo penale ormai è obiettivo improcrastinabile di questa maggioranza, finalizzato al raggiungimento di quell'efficienza che tutti gli *standard* internazionali ed europei ci impongono, dal punto di vista sia della ragionevole durata sia della certezza della pena, unitamente a un procedimento di reinserimento del reo nella società, una volta avvenuta la sua riabilitazione. La riforma del processo civile avrà come obiettivo lo snellimento delle procedure e soprattutto lo svecchiamento di istituti ormai obsoleti, utili soltanto al rallentamento del procedimento, senza allo stesso tempo ingenerare garanzie ulteriori nei confronti di chi nel processo è impegnato. la Commissione giustizia, cito i processi telematici e la giustizia telematica che, anche attraverso l'utilizzo dello strumento della PEC, renderanno le notificazioni più snelle ed efficaci; l'implementazione dell'informatizzazione degli uffici e la relativa formazione del personale; il contrasto ai cosiddetti matrimoni forzati, l'orrenda pratica purtroppo ancora molto diffusa nel mondo, un fenomeno assolutamente da stroncare;

In ambito internazionale, purtroppo, ci troviamo in un momento storico dove la minaccia globale dettata dal terrorismo rappresenta la criticità più importante da risolvere. Per questo motivo un lavoro scrupoloso, proficuo e sinergico è stato portato avanti tra i Paesi dell'Unione europea e i Paesi terzi, assicurando un rafforzamento della cooperazione giudiziaria e una presenza costante ai diversi negoziati europei e internazionali. Questa è l'azione riformatrice del Governo del cambiamento in materia di giustizia. Questo è quello che ci prefiggiamo di fare, ovvero una compiuta riforma della giustizia, che sia più in linea con la ragionevole durata dei processi e soprattutto più vicina ai cittadini: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

Chiedo ai proponenti se intendono espungere dal testo della risoluzione i punti sui quali il Governo ha espresso parere contrario e accettare le riformulazioni, nel qual caso la proposta di risoluzione nel suo complesso

Se questo lavoro è stato fatto nello spirito di lasciare agli atti di quest'Assemblea un elenco di osservazioni alla relazione del Ministro e, quindi, se decidessimo di votare per parti separate e alcune di esse sono quelle su cui il Ministro ha dato parere favorevole, possiamo considerare il voto su quella parte un'osservazione - vale per la nostra, come per le altre risoluzioni - che va a unirsi in un elenco di osservazioni che quest'Assemblea lascia agli atti?

Se l'Assemblea accetterà di votare per parti separate, non credo che il Governo cambierà il parere su quei singoli punti che lei, senatore Ferrari, mi ha indicato, perché la votazione avviene per parti separate: rimarrà favorevole su alcuni punti e contrario su altri.

così come proposto, esattamente come riteniamo di mantenere i punti sui quali il Governo ha espresso parere contrario, ovvero i punti 14) e 15).

ha sottolineato e rivendicato l'unitarietà della sua risoluzione e - dall'altro - ne chiede il voto per parti separate. Deve essere chiaro se si vota

la parola il presidente della Commissione lavori pubblici e comunicazioni, senatore Coltorti, per riferire sui lavori delle Commissioni riunite

Signor Presidente, noi, fin dall'inizio, abbiamo fatto ogni cosa che fosse nelle nostre facoltà per agevolare l'esame di questo provvedimento. Abbiamo acconsentito ieri a rinviare ad oggi. La presidente del nostro Gruppo, la senatrice Bernini, aveva già avvisato che, probabilmente, oggi ci saremmo trovati nella medesima situazione e infatti, guarda caso, questo si verifica di nuovo. Devo dire che, se

in qualche modo, più comprensibile. Il problema è che i lavori delle Commissioni sono sospesi, sono stati sospesi a lungo e, a quanto pare, resteranno sospesi. Non è che adesso chiudiamo l'Aula e le Commissioni si riuniscono: le Commissioni si riuniranno poi. Questo vuol dire che l'esame del provvedimento è stato trasferito in altra sede:

del Parlamento tutto, della maggioranza e dell'opposizione, perché la maggioranza ha presentato tanti emendamenti, addirittura più dell'opposizione, sicuramente molti interessanti, tutti rappresentativi di qualche realtà. Il fatto che si ritardi per poi comprimere l'esame tutto in un giorno solo

Non avanzo una richiesta specifica, ma chiedo che vi sia serietà e rispetto per quest'Assemblea, perché non è la prima volta. Già se fosse la prima volta sarebbe troppo, ma non è la prima volta: l'abbiamo visto sulla legge di bilancio, con riflessi persino nel messaggio di fine anno del Capo dello Stato, che poi, giustamente, è stato ripreso dal Presidente del Senato e da altre alte figure istituzionali. Ci vuole rispetto per la funzione che il Senato rappresenta. Mi permetto di dare due consigli da amico, come avrebbe detto il nostro collega della scorsa legislatura, ai colleghi della maggioranza: è normale che ci siano delle trattative all'interno della maggioranza. Succede, a volte, addirittura all'interno dello stesso partito, però, vi do due consigli. Il primo è: considerate le scadenze dell'Assemblea come vere scadenze. scadenze. Sarebbe maggiormente rispettoso delle prerogative del Senato e sarebbe più produttivo dal punto di vista delle trattative perché se alle ore 17 bisogna andare in Aula, vuol dire che alle ore 17 bisogna essere arrivati a un compromesso, a un accordo.

viene messo dentro di tutto. Non è vietato fare tanti piccoli provvedimenti; farne uno grande, per poi avere un esame così farraginoso e, addirittura, così non esistente sotto certi aspetti, nonostante il grande lavoro svolto da tutti, da entrambe le Commissioni e da tutti i colleghi che hanno partecipato ai lavori delle Commissioni, finisce per non essere produttivo. Allora, anziché infilare emendamenti di qualunque argomento su qualunque questione, a rimedio dei guai fatti nella legge di bilancio, fate dei provvedimenti diversi, di modo che si possano esaminare in modo trasparente. L'offesa non è a al Senato, ma un'offesa al Paese, Paese, che ha diritto a vedere i provvedimenti e sapere chi vota a favore e chi vota contro, non un provvedimento d'insieme, che è *omnibus* e riguarda di tutto, ma singoli provvedimenti, così come prevede la Costituzione, così come prevede il Regolamento del Senato. Ci vuole serietà per fare le cose per bene.

si rischia di rimanere senza parole, perché è l'ennesima volta che ci troviamo in una situazione, a nostro avviso, grave e di mancanza di rispetto del funzionamento dei lavori di questa Assemblea e delle prerogative di tutti i senatori. Approfitto della sua presenza, Presidente, anche per ribadire ciò che avevo avuto modo, nella sospensione di ieri mattina, di ricordare a questa

non è stato un esercizio di creatività natalizia. Lo abbiamo fatto per impedire che venissero compresse le prerogative del Parlamento e del Senato perché durante l'esame della legge di bilancio le stesse prerogative sono state profondamente lese, con un atteggiamento che rischiamo di ritrovarci esattamente negli stessi termini in questi giorni. Lo ha ricordato anche il senatore Malan: persino il Presidente della Repubblica è dovuto intervenire, dopo quello che è accaduto nel mese di dicembre, per segnalare che c'era stata una compressione dell'*iter* legislativo che è inaccettabile, al punto che la Corte ha dovuto ricordare che fatti di questa natura non sarebbero passati inosservati e difficilmente avrebbero potuto superare il vaglio di costituzionalità di lì in avanti.

Qual è il rispetto che viene portato alle opposizioni, che hanno il diritto di esaminare in profondità ogni parte del provvedimento, un diritto che hanno esercitato senza svolgere nessuna attività di ostruzionismo in queste due settimane di tentato lavoro in Commissione?

le prerogative per un relatore di maggioranza o di minoranza o per un senatore che decide di intervenire in discussione generale sono le stesse di colui che decide di intervenire in dichiarazione di voto o illustrazione di un emendamento. È quindi diritto di chi interviene in discussione generale o fa la relazione di maggioranza o di minoranza conoscere il provvedimento nella sua interezza e perché questo accada serve, questa volta, anche per agevolare il lavoro degli uffici, che ci sia un tempo adeguato tra quando vengono conclusi i lavori in Commissione e quando finalmente si incardina il provvedimento in Aula. in Aula. Siamo di fronte - e questo mi consente di richiamare il nodo politico di questa vicenda, perché poi al fondo c'è sempre un nodo politico - all'ennesima bulimia legislativa.

si producono "parti" che vanno a riempire qualsiasi provvedimento legislativo aperto. Stiamo parlando di un decreto-legge che dovrebbe rispettare il requisito dell'omogeneità di materia e se succede un fatto di attualità, si interviene, addirittura modificando il codice penale, inserendo uno modifica al codice stesso

fascicoli che non sono ancora stati chiusi; alcuni di questi, che guarda caso hanno proprio le caratteristiche che ho citato - penso al tema delicatissimo delle trivelle e alle questioni energetiche - non sono mai stati aperti e si sono già riunite due Conferenze dei Capigruppo per stabilire come discutere in Aula questo provvedimento. Lega e MoVimento 5 Stelle la smettano di continuare a lisciare il pelo al Paese, rispondendo immediatamente con il tentativo di normare tutto quello che accade nell'attualità, ed abbiano rispetto quando si assumono l'impegno di portare un provvedimento in Aula e, soprattutto, abbiano rispetto di tutti coloro che in Commissione intendono completare il lavoro discutendo fino in fondo delle questioni.

quello che varie volte ci ha indicato la Consulta, vale a dire il fatto che i decreti devono essere assolutamente omogenei e che lo stesso lavoro emendativo non può uscire dal binario dell'omogeneità.

la questione delle trivelle e le scelte energetiche. Guardate, non c'è nulla di male nel fatto che ci sia uno scontro, perché ci sono visioni diverse, ma questo deve avvenire non a lato, ma all'interno all'interno della discussione nelle Commissioni, perché io voglio discutere e non voglio soltanto dire se sono d'accordo o meno sull'emendamento su cui magari è stato già trovato l'accordo. È una

ma non possiamo più, in virtù di tutto questo continuare a rinviare, facendo in modo che le Commissioni e quindi l'Assemblea si riuniscano all'improvviso, non si sa bene con quali tempi né con quale

anche la Commissione bilancio ne ha espressi alcuni. Ci sono nodi politici, benissimo: non venite più a raccontarci le balle che tra di voi va tutto bene, sappiamo perfettamente che ci sono problemi. Ma vogliamo anche

in quest'Aula, di fronte a lei, signor Presidente del Senato, e ai senatori in base a quali leggi e Regolamenti un Ministro della Repubblica, funzionario dello Stato e generale dei Carabinieri, intenda non rispettare atti obbligatori, che la legge impone anche a lui. Vorrei capirlo dalle sue parole in quest'Aula, signor Presidente, e credo che anche lei abbia questa curiosità, come ce l'ho io: non possiamo più rimanere zitti di fronte allo spettacolo a cui purtroppo assistiamo. La maggioranza porti questo emendamento, se è il caso di farlo, altrimenti lo accantoni o lo rinvii. Faccia quello che crede, ma la nostra pazienza è terminata. È davvero terminata, Presidente, perché abbiamo atteso anche troppo. E non ci venga domani a dire che dobbiamo stare qua fino a venerdì, fino a sabato o domenica, a seconda dei comodi della maggioranza, del Ministro o del Vice Ministro, perché noi intendiamo esaminare soprattutto quell'emendamento. Vogliamo leggerlo in controluce, esaminarlo in maniera dettagliata per capire quello che dice, perché se un Ministro della Repubblica ha annunciato che si dimetterà nel caso in cui una sola trivellazione, anche già autorizzata, verrà effettuata, voglio capire se questo Ministro sarà coerente con se stesso fino alla fine, altrimenti

Ci aspettiamo serietà dal ministro Costa. Lo vogliamo domani qui in Aula e vogliamo che ripeta di fronte a noi quello che ha detto alla stampa e commenti l'emendamento che domani probabilmente, speriamo, la maggioranza sarà in grado di presentare.

delle istituzioni, del Presidente della Repubblica, del Presidente del Senato e del Parlamento, la nostra intenzione è di evitare quello che è successo anche durante la manovra economica. Proprio per questo motivo, abbiamo

Questo è il nostro intento. Chiediamo scusa se ci sono stati dei ritardi, ma che il confronto politico possa avvenire in Commissione mi sembra un po' un po' particolare. Ci può stare che ci sia un confronto su vari temi. Tra l'altro gli emendamenti sono tanti; il decreto-legge è partito con quattro articoli, ma tutti gli emendamenti che sono

necessità che il Parlamento mantenga le proprie prerogative. Intendiamo lavorare in questa direzione; se c'è la vostra collaborazione, così come c'è stata fino adesso, pensiamo davvero di poter proseguire i lavori questa sera, arrivare domani mattina in Assemblea e avere tutto il tempo necessario (visto che è programmata una seduta

per rispetto delle istituzioni, e tutto deve avvenire in modo trasparente. Se chiediamo un po' di tempo in più per un confronto su alcuni emendamenti o per alcuni pareri, penso che questo non significhi togliere prerogative al Parlamento. Questo è il nostro intento. Poi Poi sentiremo anche il collega Patuanelli e cercheremo di trovare conferma nella volontà di tutta la maggioranza di andare in questa direzione. Spero che questo possa essere sufficiente per tranquillizzare le minoranze.

il dibattito politico che si apre sui temi che vengono discussi nelle Commissioni è un dibattito spesso interessante. Ha ragione la senatrice De Petris: più spesso ci dovrebbero essere confronti politici, anche accesi, a prescindere dagli schieramenti e dalle maggioranze, in quest'Assemblea e nelle Commissioni. È chiaro, poi, che la sintesi - soprattutto per chi chi governa il Paese, quindi le forze di maggioranza - si trova prima di arrivare al voto e alle discussioni definitive sui provvedimenti.

approfondendo e analizzando nel dettaglio quei temi, e così è stato per altri argomenti. Quindi, certamente non abbiamo contratto i tempi; certamente abbiamo dato la possibilità alle opposizioni di leggere le proposte della maggioranza e alla maggioranza di valutare le proposte dell'opposizione. Diversi emendamenti dell'opposizione sono già stati accolti, all'interno dei numerosi emendamenti - credo oltre 50 - che sono stati approvati. Abbiamo votato quasi 400 emendamenti su un *corpus* emendativo che era inizialmente di 1.000

di migliorare il decreto-legge, qualche volta anche esondando dai temi del provvedimento, ragion per cui, giustamente, le Presidenze delle due Commissioni riunite hanno dichiarato talune inammissibilità, che non sono state monodirezionali, ma, come dicevo prima, equamente distribuite tra gli emendamenti, analizzandoli nel merito. Come era già evidente dagli interventi che mi hanno preceduto, la nostra proposta è quella di continuare a lavorare questa sera in Commissione, arrivare domani in Aula dopo un ampio dibattito e affrontare le undici ore che vengono garantite al dibattito parlamentare per approvare finalmente la legge di conversione del decreto-legge.

Prendo atto delle parole dei Capigruppo di maggioranza e credo che siano in assoluta buona fede. ho notato la stessa buona fede da parte del Presidente della 8a Commissione, perché non ci ha riferito esattamente sull'andamento dei lavori. È evidente, infatti - basta leggere le *news* dei tanti siti dei giornali o di informazione - che c'è un problema politico, non c'è un problema di tempi, signor Presidente. C'è un problema politico grosso, che evidentemente la maggioranza non è ancora riuscita a risolvere. Mi sembra che - in un modo garbato, in termini parlamentari - ci stiano chiedendo tempo per arrivare comunque a completare i lavori all'interno delle Commissioni riunite

Governo vara un decreto-legge vuol dire che ha dei motivi di emergenza, di urgenza. Approvando un decreto-legge si coinvolge la responsabilità della Presidenza della Repubblica, si sottopone il testo al Presidente della Repubblica. Invito, allora, il Governo a stare attento rispetto all'utilizzo del decreto-legge come un taxi per tutte le esigenze che emergano, perché non è questa la natura del decreto-legge. Signori rappresentanti del Governo, non è questa la sua natura, non è questo l'utilizzo che potete fare dei decreti-legge e non è questo l'utilizzo che il Parlamento, il Senato e la Camera dei deputati, vi può permettere di fare.

a fare i confronti di maggioranza piuttosto che a svolgere l'attività parlamentare. Troppe sono le interruzioni, i ritardi e i giorni che sono stati persi e che umiliano, ancora una volta, l'attività del Parlamento e nello specifico del Senato.

comprensione per certi tipi di atteggiamento da parte di questo Governo, della maggioranza e dei partiti che sostengono il Governo. Detto ciò, sono obbligato a chiederle la convocazione di una Conferenza però prendo atto di quanto c'è stato detto dai Capigruppo della Lega e del MoVimento 5 Stelle e reputo che sia opportuno - è un suggerimento che le do, se dovesse ritenerlo utile - convocarla per domani mattina, per vedere se la notte porterà consiglio alle forze di maggioranza, se riusciranno a trovare l'accordo sulle trivelle e a non inventarsi ulteriori temi che dovrebbero essere chiaramente esclusi

umiliazione delle Commissioni, dei parlamentari, del Senato tutto e delle nostre funzioni istituzionali. Come spesso mi sono permesso di fare, richiamo nuovamente la Presidenza a tutelare fino in fondo le nostre prerogative, i nostri diritti e i nostri doveri, che mi sembra il Governo abbia attitudine

in piazza, anche davanti al CARA, per manifestare contro questo sgombero), che questa esperienza è stata, ed è, un esempio vero di integrazione. C'erano moltissimi insegnanti, perché i bambini sono andati

In particolare, molti di questi sono già stati sgomberati dal centro e di fatto non hanno una destinazione.

un'esperienza positiva. Non si è intervenuti laddove c'erano dei problemi, ma si è intervenuti e si sta intervenendo pesantemente laddove vi è un'esperienza positiva di integrazione, di possibilità di lavoro in una comunità, perché queste persone si erano integrate nella comunità e ne sono dimostrazione le proteste

dove saranno portati i rifugiati, qual è il loro destino. In questo modo che cosa si vuol fare? Si vuole provocare un incidente? Qual Qual è l'intenzione del Ministro dell'interno? Forse sappiamo qual è l'intenzione: quella di dare lezioni, ma non è un caso - e a questo noi non ci staremo mai